La seduta è aperta

Onorevoli colleghi, si è spento ieri, a Bologna, Beniamino Andreatta. A nome del Senato della Repubblica e mio personale, desidero quest'oggi rinnovare alla moglie Giana, ai figli e ai familiari il sincero e profondo cordoglio già espresso in un messaggio appena appreso della scomparsa. Colpito da grave malore il 15 dicembre 1999 mentre seguiva, dal suo banco alla Camera, l'esame della legge finanziaria, non si è mai più ripreso e, da allora, era ricoverato all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, esemplarmente accudito dalla sua famiglia, circondato dall'affetto dei suoi cari, visitato dai suoi amici. Dopo sette anni ha dunque avuto termine questa silenziosa presenza. L'Italia perde definitivamente un suo grande figlio; sono certo dell'intenso dolore provato da tutti coloro che, come tanti di noi qui hanno avuto la fortuna di conoscerlo e incrociarlo lungo il percorso della propria esperienza umana e politica. Più volte Ministro, a lungo parlamentare, eletto al Senato (dove ricoprì anche il ruolo di Presidente della Commissione bilancio) e poi alla Camera dei deputati, la sua personalità spicca nel panorama politico italiano sin da quando, giovane professore, collabora con Aldo Moro. Nell'esercizio delle sue alte responsabilità di Governo al Bilancio, al Tesoro, agli Esteri e alla Difesa - solo per citarne alcune - si è costantemente contraddistinto per un rigore intellettuale e morale che si coniugava a una grande passione civile. Ha affrontato snodi non semplici, manifestando, accanto alla riconosciuta competenza, un costante e solido senso dello Stato e dell'interesse generale, sempre, anche quando decisioni e opinioni potevano costare l'impopolarità. Brillante economista, studioso raffinato e dotato di originalità di pensiero, inesauribile fonte di proposte e approcci per affrontare in maniera moderna e volta al futuro i grandi problemi dell'economia, dello sviluppo e della finanza del nostro Paese e convinto sostenitore dell'Europa e del valore dell'unità dei popoli europei. Beniamino Andreatta è stato anche una figura centrale nel panorama del cattolicesimo politico italiano che gli deve molto, come a poche altre personalità nella nostra storia. Maestro di tantissimi giovani, non solo nell'università, ma anche nella politica, aveva saputo, anche per questa strada, dare un'indicazione precisa e inequivoca: il futuro del Paese, di ogni Paese, è nelle mani dei giovani, a cui le generazioni che li hanno preceduti devono, con generosità, trasferire con le competenze la fiducia e la voglia di andare più avanti. Credo sia giusto dedicare quanto prima una riflessione dell'Aula a Beniamino Andreatta, al suo forte impegno parlamentare e al grande contributo di pensiero che ha fornito all'Italia durante tutta la sua vita. *(Generali applausi)*. Vi invito ad osservare un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, desidero aggiungere solo poche parole al ricordo di Beniamino Andreatta e, in modo particolare, da lui svolta, qui in Senato, come Presidente della Commissione bilancio. In un momento particolarmente difficile e di grande turbolenza interna democratico-cristiana, dovemmo al suo equilibrio e alla sua dedizione il superamento, senza troppi guai, di quella circostanza. Vorrei aggiungere che anche

Grazie,

apre una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 aprile. Oggi pomeriggio, come già stabilito, proseguirà la discussione del decreto-legge recante proroga di missioni internazionali, fino alla votazione finale. Le dichiarazioni di voto - per le quali sono stati attribuiti a ciascun Gruppo dieci minuti aggiuntivi (quindici al Gruppo misto) rispetto ai tempi già consumati - avranno inizio intorno alle ore 19. E' pervenuta dal prescritto numero di senatori richiesta di remissione all'Assemblea del parere della 1a Commissione permanente sui presupposti di costituzionalità relativi al decreto-legge in materia di liberalizzazioni. La deliberazione sui presupposti di costituzionalità è stata posta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani. Esaurita tale fase procedurale, la seduta dell'Assemblea sarà tolta per consentire la convocazione delle Commissioni, in particolare della 10a Commissione permanente e delle altre Commissioni impegnate nell'esame del decreto-legge sulle liberalizzazioni, che pertanto avranno a disposizione tutta la parte residua della giornata di domani. La discussione del decreto in Assemblea, in relazione al termine di scadenza, avrà inizio nella seduta antimeridiana di giovedì 29 marzo con prosieguo nella giornata di venerdì 30. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi. Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, resta confermato nel pomeriggio di martedì 3 aprile, previa ripartizione dei tempi tra i Gruppi, l'esame del decreto-legge sulla violenza nelle competizioni calcistiche, ove modificato dalla Camera dei deputati. La discussione del bilancio interno e dei rendiconti consuntivi del Senato avranno luogo nella seduta antimeridiana di mercoledì 4. Il calendario della settimana prima di Pasqua prevede inoltre le mozioni sull'industria agroalimentare e la mozione Bianconi sulla medicina di genere. Nella settimana dopo Pasqua l'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 11 e giovedì 12 aprile per l'esame di ratifiche di accordi internazionali, delle mozioni eventualmente non concluse, della mozione Schifani ed altri sull'annullamento del decreto ministeriale sull'uso personale di stupefacenti, nonché del disegno di legge delega per il riordino degli enti di ricerca.

di scienza, di cultura, di onestà intellettuale Beniamino Andreatta. Egli ha dato lustro a quest'Aula, al Governo italiano. Ho convissuto con lui momenti anche difficili come collaboratore. Abbiamo trascorso nottate di dibattito sul piano della politica economica e sociale del Paese. Non mi dilungo oltre, perché l'emozione prevale rispetto a ciò che sarebbe dovuto a Beniamino Andreatta per quello che ha dato al nostro Paese. Debbo aggiungere un ringraziamento personale per trentacinque anni di convivenza, anche, nell'ultimo periodo, con differenze di opinioni tra noi, ma sempre con una grande, reciproca

Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali,

esprimerò i pareri sugli ordini del giorno da G1 a G7; G7; il relatore per la Commissione affari esteri, senatore Tonini, esprimerà poi i pareri sugli ordini del giorno da G8 a G14. È appena il caso di aggiungere che questa suddivisione del nostro lavoro riguarda la prevalenza delle materie trattate in ciascun ordine del giorno e e che quanto diremo è totalmente condiviso da entrambi i relatori. Cominciamo dagli ordini del giorno G1, a firma Calderoli,

Questi ordini del giorno concernono, sia pure in termini differenziati, un argomento comune a tutti e tre, ossia l'esigenza di dotare il contingente militare italiano in Afghanistan degli strumenti e degli armamenti idonei a far fronte ad una situazione di crescente gravità. Mi sia consentito richiamare all'attenzione dei signori senatori che, in sede di replica alla discussione generale sul provvedimento, fu sottolineata dai relatori la raccomandazione al Governo affinché, nell'ambito degli accordi che regolano la partecipazione italiana alla missione ISAF, si provveda ad ogni dotazione di mezzi e di armamenti che si renda utile alla sicurezza dei militari e dei civili italiani presenti in Afghanistan, alla protezione della popolazione ad essi affidata e al pieno svolgimento della missione secondo il mandato ricevuto fin dal 2001 dalle Nazioni Unite. Nella sua replica in quest'Aula, nella seduta notturna che lei ha richiamato poc'anzi, venne dal Governo la piena conferma della volontà, della determinazione di assicurare al contingente italiano gli assetti necessari in termini di *intelligence*, di armamenti e di mezzi, in modo da consentire il pieno controllo del territorio e la prosecuzione della missione con la massima sicurezza sia per i militari, sia per i civili operanti in Afghanistan. Dunque, in questa materia sussistono - se la considerazione non è di troppo ottimismo - ragioni sufficienti per riscuotere in quest'Aula una larga convergenza di opinioni e di voto.

che possa valere ad ottenere il ritiro di questi tre ordini del giorno e la convergenza su una comune opinione. Non voglio tuttavia sottrarmi all'obbligo, che compete al relatore, di pronunciarsi circa il voto che, nel caso i tre ordini del giorno fossero portati alla votazione dell'Assemblea, dovrebbe, a nostro avviso, orientarla.

il dispositivo è accettabile in quanto in larga parte analogo a quello dell'ordine del giorno precedente; non sono accettabili invece le motivazioni in premessa, in cui si esprimono a carico della condizione attuale della nostra missione in Afghanistan valutazioni negative che, a nostro avviso, non trovano oggettivo fondamento.

contenute nella premessa e nelle considerazioni si associano in maniera difficilmente separabile dallo stesso dispositivo. del giorno, che abbiamo potuto vedere soltanto in questi minuti, contiene poi una serie di specificazioni circa nuovi, ulteriori, sistemi d'arma di cui si dovrebbe dotare il nostro contingente in Afghanistan che, a nostro avviso, meglio competono alla responsabilità degli stati maggiori. Pertanto, confidando che quanto dirà tra poco il Governo valga ad ottenere il consenso ampio dell'Assemblea

I successivi ordini del giorno G2 e G3, entrambi a firma del senatore Calderoli, saranno anch'essi oggetto, io credo, di una specifica e precisa proposta da parte del Governo e dunque, a maggior ragione, anche rispetto ai precedenti, converrebbe considerare la possibilità di ritirarli. l'ordine del giorno G2 impegna il Governo ad escludere la partecipazione ad un'eventuale Conferenza internazionale di pace di rappresentanti di forze belligeranti che non abbiano deposto le armi. Forse è un eccessivo scrupolo formalistico osservare che siccome l'eventuale Conferenza di pace non sarà organizzata dal Governo italiano, bensì dalle Nazioni Unite, converrebbe comunque dire che si chiede al Governo di adoperarsi per escludere e non di escludere direttamente, cosa che non sarebbe nei suoi compiti. certamente evidente che la rinuncia allo stato di belligeranza e all'uso delle armi è precondizione necessaria per una conferenza di pacificazione.

Qualora si arrivasse al voto su questi due ordini del giorno, salva, come si auspica, la possibilità di trovare un'intesa sulla base delle precise proposte che il Governo potrà formulare in proposito, il proposito, il parere dei relatori su entrambi è negativo. L'ordine del giorno G6 è stato presentato dal presidente Cossiga,

questa è una fase in cui ci sono moltissimi senatori che vogliono seguire con serietà il relatore. Non è ammissibile questo mormorio che impedisce ai colleghi di seguire con attenzione e disturba il relatore.

che sia soprattutto accettata dalle popolazioni civili, delle associazioni democratiche e della società civile afghana, lavorando al contempo alla possibilità di una trasformazione della presenza internazionale nel Paese», sopprimendo le tre righe seguenti. nel paese; «» *b)* sostenere processi di giustizia di transizione e di riconciliazione nazionale contribuendo alla formazione di una Commissione indipendente per la verità e la giustizia che faccia chiarezza sui crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani;

«impegna il Governo a riferire alle Camere con cadenza trimestrale, più ravvicinata quindi da quella già prevista nel decreto, in ordine ai cambiamenti e/o integrazioni del ruolo e del senso della nostra missione in Afghanistan». Come relatori, ci siamo sempre dichiarati favorevoli a tutte le proposte che vadano nel senso di un monitoraggio più stringente di tutte le nostre missioni.

Invito i colleghi a prestare particolare attenzione a questo ordine del giorno che tratta una materia particolarmente delicata, come quella riguardante la gestione degli episodi di sequestri di persona a scopo di terrorismo.

con il più intimo e delicato degli *arcana imperii* - per così dire - che dovrebbe essere lasciato al Governo. Naturalmente, ci sono leggi e regole internazionali che il nostro e gli altri Governi sono tenuti ad osservare; nell'ambito di queste regole e criteri credo sia indispensabile, per questo come per qualunque Governo della nostra Repubblica,

vorrei - se mi è consentito - affrontare alcune questioni perché devo anche motivare delle proposte, nella speranza che possano trovare accoglimento, anche perché il Governo è sensibile - voglio dirlo subito - ad alcune questioni che sono poste negli ordini del giorno che sono all'esame del Senato. il Governo è sensibile all'esigenza sollevata, in alcuni ordini del giorno, di fornire i nostri militari di mezzi adeguati per la protezione del personale militare e civile in relazione a un'aumentata pericolosità delle condizioni in cui opera il nostro contingente. Vorrei, da questo punto di vista, informare il Senato che i Ministeri e i Ministri della difesa e degli esteri hanno incontrato, giovedì scorso, lo Stato Maggiore delle Forze armate italiane

pervenire al più presto al Governo una relazione che indichi anche le condizioni che le Forze armate ritengono indispensabili alla protezione del personale italiano, alla protezione dei civili afghani che sono affidati alla protezione del personale italiano in relazione alla situazione in atto nelle province e nelle aree di nostra competenza. Vorrei, quindi, rassicurare il Senato che il Governo ovviamente intende provvedere e provvederà, previa informazione delle Commissioni competenti, sulla base di una relazione tecnica che sia predisposta dallo Stato Maggiore delle Forze armate, che credo meglio di noi possa valutare le necessità dal punto di vista tecnico di protezione dei nostri militari. Lo dico perché appunto non è a noi estranea la preoccupazione che ha mosso diversi parlamentari e perché abbiamo già avviato una procedura per dare a questa preoccupazione una risposta efficace, previa ovviamente l'informazione del Parlamento; qualora queste necessità operative comportassero nuove misure di finanziamento, il Governo vi provvederà *ad hoc*. Vorrei anche dire naturalmente, perché nei giorni scorsi si è sviluppata un'appassionata discussione nella quale in molti momenti non è parsa chiara la distinzione tra regole di ingaggio, *caveat* e attrezzature dei nostri militari, che naturalmente il dotare i nostri militari di mezzi più adeguati alla loro protezione non significa mutare la natura della missione; né le regole di ingaggio sono nelle nostre disponibilità perché, com'è noto, sono decise da chi ha la responsabilità della missione militare (la NATO e le Nazioni Unite). Per quanto riguarda i *caveat*, essi riguardano, com'è noto, la disponibilità delle Forze armate italiane nelle aree che ci sono state assegnate e il Governo ha già spiegato che non intende rimuovere queste limitazioni.

impegnare il Governo a fornire al contingente italiano in Afghanistan, ferma restando la natura della missione, i mezzi necessari per una più adeguata protezione del nostro personale militare e civile sulla base della aggiornata valutazione dello Stato Maggiore, previa informazione alle competenti Commissioni parlamentari. Se questo ordine del giorno venisse accolto in tale formulazione, io esprimerei ovviamente un parere favorevole a nome del Governo, pregando di ritirare gli altri ordini del giorno sulla stessa materia che, animati da una intenzione che ci è comune, tuttavia mi appaiono ultronei, soprattutto perché già definiscono di quali mezzi dovrebbe trattarsi. Ho rassicurato il Senato che se ne discuterà sulla base di una relazione dello Stato Maggiore delle Forze armate.

e che, tuttavia, il Governo italiano ha già proposto, in particolare nella seduta del 20 marzo ultimo scorso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con una formulazione precisa che è all'esame della stessa ONU. Senza nulla togliere al valore del dibattito politico, tuttavia, quando si parla di una Conferenza internazionale per la pace proposta dal Governo italiano ci si deve necessariamente riferire a ciò che il Governo italiano ha proposto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nella seduta del 20 marzo, che è la proposta all'esame delle Nazioni Unite a cui si chiede di copromuovere la Conferenza insieme alla Germania, che, nella sua qualità di Presidente di turno del G8, presiede un organismo internazionale,

su chi dovrebbe o non dovrebbe intervenire con atti d'indirizzo parlamentare che impegnano il Governo a compiere atti che non può fare. In particolare, la nostra proposta è volta a sostenere, anche attraverso una Conferenza internazionale, quello che è stato definito il Piano per la pace e la riconciliazione nazionale in Afghanistan e vorrei ricordare a tutti noi che, al di là delle considerazioni politiche, è il Governo afghano che ha invitato al tavolo della riconciliazione nazionale le forze in campo, sia i signori della guerra, sia i cosiddetti talebani, proponendo anche all'esame del Parlamento afghano un'amnistia per i crimini compiuti nel corso del conflitto volta a favorire un processo di riconciliazione nazionale. È evidente che tale iniziativa di riconciliazione nazionale afghana è condotta dal Governo afghano e la comunità internazionale la sostiene e la incoraggia, ma non è che può sostituirsi al Governo afgano nel promuovere tale processo

il Senato, preso atto della proposta avanzata dal Governo italiano nella seduta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 20 marzo scorso per una Conferenza internazionale per la pace in Afghanistan, impegna il Governo a continuare nella sua iniziativa per una Conferenza volta, in particolare, a rilanciare l'impegno economico, sociale e civile dell'intera comunità internazionale, a promuovere una più stretta cooperazione fra i Paesi della regione e a sostenere l'impegno di riconciliazione nazionale afgano lanciato dal Governo Karzai. Poi su chi sarà invitato decideranno appunto loro, questo è naturale perché non spetta a noi deciderlo. Da ultimo vorrei rivolgere una preghiera, una richiesta al senatore Calderoli a proposito dell'ordine del giorno dell'ordine del giorno G14, che tratta della questione degli ostaggi. Si tratta di una questione estremamente delicata, com'è evidente. Certamente, la linea condotta dal Governo in occasione del rapimento del giornalista Mastrogiacomo fu diversa rispetto a quella tenuta in occasione del rapimento Moro, ma non dissimile da quella tenuta in occasioni più recenti

se si vuole andare a fondo di questa questione si deve fare un'altra cosa: si deve proporre una Commissione d'inchiesta che esamini fino in fondo il modo in cui sono state trattate tali vicende e accerti eventuali responsabilità, il Parlamento ha il potere per farlo, ma se si vuole affrontare questa questione, così

che significa esporre a rischio cittadini italiani, si riferisca esclusivamente al teatro dell'Afghanistan o valga universalmente. Ora, io ritengo che nessun Governo al mondo, nessun Paese si lega le mani in questo modo, potrei citare infiniti casi di altri Paesi che hanno negoziato per salvare la vita di loro concittadini e ritengo che la questione sia così delicata che

sede NATO, norme di comportamento comune, dato che lì siamo impegnati in una missione insieme ad altri Paesi. Più in generale, io credo che fatti di questo genere debbano essere esaminati caso per caso, a seconda dei Paesi in cui accadono e a seconda delle circostanze concrete. Ritengo che un principio generale come quello espresso in modo così semplicistico in questo ordine del giorno sia rischioso e credo che non sia giusto nei confronti di tanti cittadini italiani, giornalisti ma anche lavoratori e militari, impegnati in tante parti del mondo, ai quali noi non possiamo dire che qualsiasi cosa vi succeda, da ora in poi il Governo e lo Stato italiano se ne lavano le mani. Credo, e vi prego davvero, che una questione così delicata debba essere approfondita e discussa meglio prima di arrivare a deliberazioni così semplicistiche e universali. Pertanto pregherei

evidentemente, mi ero distratto e credevo che mercoledì scorso fossero state esaurite la discussione generale e le repliche del Governo e che oggi qui avremmo esaminato gli emendamenti e gli ordini del giorno.

il Ministro formalizzasse la prima parte del suo intervento, per cercare di capire cosa vuol dire e dove vuole andare a parare. Poi vorrei che ci riferisse cosa è accaduto, da mercoledì ad oggi, per cambiare così radicalmente l'atteggiamento del Governo attraverso questo intervento. Infatti, egli non si è limitato ad esprimere un parere, bensì è entrato nel merito e ha detto cose diverse riaprendo la discussione. Pare che sia accaduto qualcosa di così importante in queste ore, da aver fatto cambiare idea al Governo: ce lo dica molto chiaramente, in modo che ci possiamo adeguare. Altrimenti, chiedo che vi sia una sospensione, magari di un quarto d'ora, per poter esaminare i testi che il Governo vuol presentare, per vedere se sono in sintonia

non riesco a capire come possa il Governo pensare che possiamo ritirarli a fronte di una promessa vaga e fumosa, senza alcun impegno. Ricordo, infatti, che gli ordini del giorno già sono di secondo rango, perché sono cogenti semplicemente dal punto di vista

Signor Presidente, credo che il collega Matteoli abbia detto una cosa molto utile, perché il ministro D'Alema ha mostrato di esprimere un parere a suo giudizio conclusivo sull'intera questione posta dai diversi ordini del giorno, che riguardano genericamente il rafforzamento delle nostre Forze armate.

Senatore Selva, ha già preso la parola il suo Capogruppo. Ora stiamo vedendo di chiarire un punto procedurale, poi, nel merito, potrà parlare. Resto ancora dell'avviso che gli ordini del giorno sono questi. Sono state fatte alcune considerazioni che non toccano la responsabilità dei presentatori, che poi possono intervenire e decidere ciò che vogliono fare nel dibattito.

Stiamo a questo punto. Quindi, pregherei i colleghi di procedere allo svolgimento ordinario dei nostri lavori. Siamo d'accordo secondo le indicazioni date dal senatore Castelli?

Signor Presidente, non sono riuscito a leggere il Regolamento del Senato, ma, riferendomi a ciò che accade alla Camera, quando nel corso del dibattito un Ministro prende la parola, come è stato il caso del ministro degli affari esteri D'Alema, che ha parlato anche a nome del Ministro della difesa - anzi, a questo proposito, apro una parentesi, c'è un illustre sconosciuto nel nostro dibattito, il Ministro della difesa, che non si è mai presentato in quest'Aula quando si parla di militari.

Ho qui la proposta di riformulazione - quindi, siamo sempre sui singoli ordini del giorno

che è emersa una novità politica significativa. Cioè, le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri rappresentano una novità politica significativa sulla quale egli chiede di avere il tempo di fare una riflessione

cambiamento significativo di una posizione politica. Se si chiede tempo per riflettere, vuol dire che c'è qualcosa su cui riflettere. Non capisco perché debba essere impedito un atto di civiltà la dimostrazione che c'è una volontà di capire e di riflettere. Questo può portare ad instaurare in Parlamento un miglior dialogo fra maggioranza e opposizione. Perché dire di no?

proponesse un ordine del giorno o una risoluzione. Di solito, sono i Gruppi a farlo, non il Governo a presentare un ordine del giorno rivolto a se stesso. Evidentemente, il Governo ha cercato di recuperare qualche ordine del giorno che non era stato presentato. avviso, con le risoluzioni e con gli ordini del giorno non si può risolvere il problema, mi permetto di proporre al Governo, l'unico che lo può fare al punto in cui siamo arrivati,

«A seguito della richiesta dello Stato maggiore della difesa, il Governo dispone l'immediato adeguamento delle dotazioni in armamenti, mezzi e tecnologie al fine di garantire sia le condizioni di massima sicurezza del personale impiegato, sia la più efficace collaborazione con le altre forze dell'ONU presenti sul campo». Se il Governo accetta di presentare questa modifica,

e stiamo discutendo ordini del giorno presentati dall'opposizione. Sentiamo ora dalle parole dell'amico Matteoli che gli ordini del giorno non servono a nulla, ragion per cui ci si domanda a quale scopo essi siano stati sottoposti all'esame di quest'Aula così importante. vorrei rispondere: noi stiamo discutendo gli ordini del giorno. Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G1, esattamente come è nei poteri del Governo e nella prassi parlamentare. Non ha proposto una risoluzione, né altro. Perché il Governo ha proposto una riformulazione? Perché diversi ordini del giorno, in modo del tutto appropriato, si pongono il problema di assicurare ai nostri militari i mezzi idonei alla protezione del personale militare e civile e dei civili afgani che vivono nelle aree a noi assegnate dalla missione delle Nazioni Unite. Il Governo intende farsi carico di questa esigenza e per l'impegno congiunto del Governo, del Ministero della difesa, del Governo nel suo insieme, io ho informato il Senato che abbiamo già avviato la procedura per ottenere dallo Stato maggiore delle nostre Forze armate un'indicazione dettagliata dei mezzi ritenuti necessari per la protezione dei nostri militari. Ho anche detto al Senato che non appena questa relazione sarà disponibile il Governo informerà le Commissioni competenti e provvederà a fornire il nostro contingente di questi mezzi: è una dichiarazione seria, solenne, verificabile, perché nei prossimi giorni questo sarà all'esame di tutti. giorni questo sarà all'esame di tutti. Noi stiamo discutendo un decreto di finanziamento, non una legge delega o un provvedimento programmatico: tradurre in un emendamento un provvedimento il cui contenuto ad oggi ci è ignoto, perché noi dobbiamo finanziare l'impiego di mezzi determinati e lo faremo sulla base di una relazione tecnica, a mio giudizio (lo dico onestamente, essendo mosso dalle intenzioni di un dialogo sereno e non strumentale) non è possibile ed è oltre tutto rischioso per un provvedimento che scade il 2 aprile, in una situazione in cui la Camera è nel pieno svolgimento dei suoi lavori con un'agenda molto fitta e complessa. Allora, se vogliamo dare una risposta a delle esigenze, il Governo è qui per assumersi le proprie responsabilità e per assumere i propri impegni nella sede della discussione sugli ordini del giorno, che è quella che stiamo facendo, non è stata una mia iniziativa. Poi ognuno sarà libero di votare come vuole sul decreto e si prenderà la responsabilità che crede; ma adesso io torno a rivolgere la mia preghiera al primo presentatore di ordine del giorno: se venisse accolto l'invito alla riformulazione fatto dal Governo, credo che potrebbe esserci un largo voto del Senato che impegnerebbe il Governo, che sarebbe ben lieto di essere impegnato, a presentarsi in un tempo rapido per chiarire quali misure ulteriori verranno prese per la sicurezza dei nostri militari. Questo se si ha a cuore il tema. Altre esigenze di natura politica, tendenti a prolungare una schermaglia anche per giustificare decisioni comunque legittime sono esigenze legittime, ma, vorrei essere chiaro, nulla hanno a che fare con il problema della protezione dei nostri militari.

in ordine al fatto che si stiano discutendo gli ordini del giorno e che la richiesta del collega Matteoli, che mi accingevo a fare anch'io sullo stesso testo, fosse fuori luogo. Vorrei spiegare che, nel momento in cui si è conclusa la fase emendativa del decreto, lo scenario del teatro afgano era - secondo noi - diverso rispetto a quello odierno,

l'attenzione è mutata e postula secondo noi un intervento normativo più stringente e vincolante, più precettivo per il Governo rispetto all'esigenza di tutelare i nostri militari. Ecco la mia risposta al ministro D'Alema in relazione alla sua acuta osservazione, là dove sostiene che si sta parlando di ordini del giorno sul tema della sicurezza: lo si fa, Ministro, perché dieci giorni fa lo scenario che analizzavamo era diverso da quello attuale. Posso assicurare al Ministro che, se lo scenario fosse stato quello di oggi, noi saremmo intervenuti con una proposta emendativa del testo del Governo e non con ordini del giorno.

del dibattito, noi sottoscriviamo la proposta del collega Matteoli. Non c'è dubbio che le dichiarazioni del ministro D'Alema, che viene ad annunciare all'Aula aver convocato, qualche giorno fa, gli Stati Maggiori dell'Esercito perché gli indichino ciò di cui adesso i nostri militari necessitano per poter operare in piena sicurezza, danno innanzi tutto

a sinistra si dà assicurazione che non si invierà un militare in più, un fucile in più o un armamento in più. Pertanto, nel momento in cui si afferma che il Parlamento per la prima volta ha dato un *input* che scuote il Ministro della difesa ed il Ministro

Mi sembra che l'ordine del giorno G1 sia di una semplicità e di una linearità assolute giacché «impegna il Governo a promuovere tutte le iniziative finalizzate a garantire la sicurezza del nostro personale militare e civile presente sul territorio afghano».

il considerando, perché è il nocciolo della questione. La necessità di adeguare gli armamenti, i mezzi e le armi difensive per i nostri soldati deriva da una necessità ben precisa e deriva proprio da quanto é stato illustrato nel considerando. Il relatore mi perdoni - forse c'era un po' di confusione prima perché c'era un'Aula abbastanza chiassosa - ma non sono riuscito a recepire come mai ha dato parere contrario al considerando, perché vi sono scritte delle cose totalmente banali,

Dopo quello che è successo al giornalista Mastrogiacomo credo sia necessario. Voglio ricordare - e su questo il ministro D'Alema potrà non fare altro che darmi ragione - che oggi i nostri

a condizioni di difesa quali quelle irachene, perché è del tutto evidente che l'evoluzione del quadro sta andando verso quella direzione. Quindi, non si riesce a capire come mai

ritengono che probabilmente i talebani aumenteranno l'offensiva? Mi spieghino, il relatore e il Governo, dove sono le parti non condivisibili di questo considerando, perché francamente non lo capisco.

non vi erano stati gli attentati e la vicenda Mastrogiacomo non aveva determinato lo scenario politico in quel teatro di guerra che ha causato una perdita di credibilità e quasi una criticità da parte di tutti gli alleati nei confronti del nostro Paese.

le nostre armi da difesa passiva a difesa attiva. Questo non significa che si va alla guerra ma significa indicare seriamente, in maniera più scientifica, di merito, di che cosa le nostre truppe devono munirsi per evitare che determinati attacchi da parte dei talebani possano trasformarsi in momenti conflittualmente pericolosi. Abbiamo voluto recepire, tra l'altro,

mezzi. Ci siamo posti, quindi, in piena sintonia con una esigenza seria che ha voluto anche andare a scavare nella metodologia e nella tipicità delle armi di cui necessitano i nostri militari.

Non c'è bisogno di sentire di cosa hanno bisogno i nostri generali: l'ha già detto, *apertis verbis,* il generale Satta l'altro giorno su uno dei principali quotidiani italiani. Egli ha dichiarato che c'è bisogno di elicotteri e di mezzi blindati, più blindati di quelli che hanno oggi i quali non sono in grado di difendersi dall'assalto dei razzi, che sono poi quelli che si portano a spalla e che quindi qualsiasi guerrigliero può avere. avere. Noi abbiamo tradotto, semplicemente e immediatamente, in questo ordine del giorno le necessità che ci sono state trasferite dal nostro esercito. Se il Governo volesse approvare questo ordine del giorno come ha dichiarato di voler approvare le richieste dei militari, potrebbe agire fin da subito e potrebbe colmare un vuoto che altrimenti sarebbe di molti giorni nei quali non si sa cosa può succedere. Colleghi, perché vi assumete questa responsabilità?

AN).* Siamo qui per discutere, non affidiamoci allo stellone, siamo noi che possiamo decidere e siamo noi che stiamo decidendo della sicurezza dei nostri ragazzi che abbiamo mandato laggiù. Non teniamoli allo sbaraglio, questo è il dato: pensateci! pensateci! Non pensate soltanto alle bandiere della pace che tutti quanti avete nascosto, tanto che non se ne vede più neanche una in giro, dove le avete messe le bandiere della pace?

Signor Presidente, onorevole Ministro, innanzi tutto vorrei ricordare al ministro D'Alema che certi impedimenti tecnici o procedurali che ha avanzato erano presenti anche durante il Governo Berlusconi, seguito di una richiesta dell'opposizione, che chiese lo spacchettamento del decreto con il quale si rinnovavano le missioni internazionali, noi spacchettammo il decreto in una notte

un metodo e una procedura che si possono sempre superare. Questo decreto, è vero, scade il 31 marzo, ma se noi lo votassimo questa sera resterebbero ancora quattro giorni alla Camera: in quattro giorni si può abbondantemente approvare, in terza lettura, il provvedimento. Entrando nel merito dell'ordine del giorno G5, che è stato firmato anche dal nostro Capogruppo, signor Ministro, le preoccupazioni sono nate nel tempo e anche per noi sono mutate le condizioni. Lei ha citato un incontro con i Capi di Stato Maggiore per conoscerne le esigenze. Io le ricordo, ad esempio, che esiste un impegno già assunto dal Governo italiano, per inviare in Afghanistan due aerei *Predator* - che non sono due aerei cattivi, come qualcuno di Rifondazione Comunista ha obiettato, non sono, cioè, strumenti di guerra solo per il nome che hanno che non sono ancora arrivati in Afghanistan. Durante il dibattito, abbiamo appreso che probabilmente arriveranno tra la fine di aprile e la metà di maggio. Lei ci consentirà di essere un po' preoccupati di questi tempi lunghi. Se due mezzi che abbiamo garantito in sede NATO dovranno arrivare in Afghanistan tra due mesi, allora l'affermazione che gli ordini del giorno hanno un peso relativo come impegno al Governo si lega al fatto che neppure impegni presi dal Governo in sede multilaterale e multinazionale corrispondono poi operativamente a ciò che deve essere fatto. fatto. Entrando nel merito dell'ordine del giorno G5, noi stiamo parlando di due *caveat* che furono scelti nel 2003 e che riguardano la provincia di Herat e la zona di Kabul. Nella provincia di Herat, voglio ricordarlo anche ai colleghi perché altrimenti il discorso diventa estremamente complicato, noi abbiamo mandato 1.000 uomini a garantire stabilità e sicurezza sul territorio in una fase nella quale, attraverso un piano di ricostruzione territoriale, la parte della cooperazione civile e della ricostruzione sembrava al momento prioritaria. È quindi ovvio che le truppe sono attrezzate ed operano per la missione che avevano nel momento in cui fu immaginata questa operazione. Oggi, anche per dire dello stesso ministro D'Alema, le condizioni sono mutate, cioè non siamo più in condizioni di garantire solo un ordine pubblico e una lotta alla criminalità organizzata e ci troviamo di fronte ad un pericolo, chiamiamolo militare.

Nel nostro ordine del giorno, peraltro, in maniera magari un po' sibillina, c'è un secondo impegno che chiediamo al Governo. Al di là del rafforzamento delle misure di sicurezza e quindi di una maggiore garanzia per i nostri militari impegnati in Afghanistan,

ma è anche curioso che, nell'ambito di questa alleanza, a mutate condizioni, ci si metta nella situazione di dire «alcuni rischi siamo in grado di assumerli, altri ve li assumete voi». Non voglio invocare la dignità nazionale, ma credo che sia un altro motivo di riflessione comprendere che i nostri militari, in un quadro multilaterale, devono essere messi nelle condizioni di operare come tutti gli altri contingenti operanti sul territorio dell'Afghanistan.

e porterà le opposizioni ad assumere un atteggiamento complessivo che magari non avrebbero voluto assumere in sede di votazione finale.

È un dato di fatto, quindi, che contraddice una parte della premessa. In secondo luogo, è stato sufficientemente chiaro il ministro D'Alema nel momento in cui ha raccomandato al Parlamento di non sostituirsi alla competenza e alla professionalità delle Forze armate che saranno, quelle sì, in grado di effettuare una ricognizione dettagliata e puntuale delle esigenze di nuovi armamenti necessari ai nostri soldati che operano in Afghanistan. In questo senso, il

Questo è un calcolo molto triste da fare e voglio soltanto dare una notizia. Nel momento in cui il Governo Berlusconi autorizzava la missione in Afghanistan, il nostro esercito ha subito in quel Paese cinque perdite e un certo numero di feriti. sono stati in quell'occasione nessun rafforzamento dei mezzi militari e nessuna strumentalità da parte dell'opposizione, mentre voglio ricordare che proprio in questi giorni abbiamo avuto soltanto un ferito lieve e questo testimonia peraltro della validità dei mezzi che, sin da settembre, il Governo Prodi ha inviato in quel teatro. Sono queste le ragioni essenziali sulla base delle quali motiviamo la nostra contrarietà

messo a disposizione del Parlamento, nel pieno esercizio delle sue prerogative e in osservanza del Regolamento, un ordine del giorno che tentava di rispondere alle esigenze poste da tre ordini del giorno, ma il relatore prima e il ministro D'Alema dopo avevano, sin dall'inizio, annunciato che in ogni caso sarebbero stati favorevoli e al primo ordine del giorno a firma Calderoli e al dispositivo del secondo ordine del giorno. Speculare anche sulla circostanza che il Senato della Repubblica abbia votato all'unanimità per il rafforzamento delle misure a tutela dei nostri soldati, francamente non mi sembra né un buon servizio alla politica, nè tantomeno un buon servizio ai nostri militari.

testo 2** Il Senato, impegna il Governo ad escludere la partecipazione ad una eventuale conferenza internazionale di pace di rappresentanti di forze belligeranti che non abbiano deposto le armi. che è un po' difficile immaginare una Conferenza internazionale di pace a cui partecipino belligeranti in armi, questo ordine del giorno può essere accettato sulla base del comune buon senso. *(Applausi

che io apprezzo nei suoi atteggiamenti in Commissione, egli ha espresso parere favorevole sulla parte conclusiva dell'ordine del giorno G8, a firma mia e di altri colleghi.

le premesse, lo svolgimento dell'ordine del giorno e le conclusioni del medesimo. L'ordine del giorno è composto non per parti separate e anche distinte. Rappresenta un'articolazione

Se la conclusione è la sintesi e la rappresentazione di tutto il contenuto del dispositivo, è un atto arbitrario che si voti per parti separate. Chiedo, personalmente, che l'ordine del giorno G8 si voti nella sua interezza.

Il Senato, preso atto delle dichiarazioni odierne del Segretario Generale della NATO, Jaap de Hoop Scheffer, in relazione al rapimento del giornalista Mastrogiacomo secondo le quali "l'azione di un singolo Paese può avere implicazioni sugli altri Paesi e può costituire un incentivo per ulteriori azioni del genere" e che il Segretario si è impegnato affinché abbia luogo una discussione a riguardo,,

trovo discutibile la definizione di «soluzione semplicistica» data dal Ministro rispetto alla mia soluzione, perché essa è la stessa con cui una legge dello Stato del 1991, la n. 82, ha fissato la linea che deve essere tenuta nel caso di sequestro. È quindi tutt'altro che semplicistica,

del Segretario generale della NATO. sgombrare il campo da un equivoco che ormai ricorre nei commenti giornalistici e anche negli interventi dei colleghi. Il blocco dei beni, cui si riferisce il senatore Calderoli, in caso di sequestro, non si applica, secondo il nostro codice penale, al caso di sequestro per scopo di terrorismo. Vorrei essere chiara.

e il Governo ad accettarlo, così come modificato, insieme al relatore, ritengo che la difesa della vita dei nostri connazionali sia un elemento di sovranità nazionale non condivisibile in nessuna alleanza e in nessuna organizzazione. Non vorrei che gli americani decidessero della vita dei nostri soldati o dei nostri rapiti all'estero, così come non vorrei che noi decidessimo della sorte di soldati o di civili americani dove si svolgono missioni NATO. Voterò quindi contro l'ordine

non mi sembra convincente. Non riesco a capire qual è la differenza tra il valore della vita di un sequestrato per ottenere del denaro e quella di un sequestrato per motivi di terrorismo politico. *(Applausi dai in quest'Aula che al tempo delle Brigate rosse enormi e terribili sacrifici sono stati fatti per difendere il prestigio dello Stato, l'autorità dello Stato e la vita dei servitori dello Stato, messa in pericolo da trattative affrettate che rimettono in libertà terroristi che tornano ad uccidere.

Presidente, ritengo che il Governo abbia operato bene per la liberazione degli ostaggi e dovrebbe continuare in questa direzione riguardo a chi si trova ancora in una situazione

intervengo sull'ordine dei lavori, ma, in realtà, per rinnovare un appello al relatore e al Governo. Noi siamo dinanzi ad una pericolosa evoluzione della minaccia talebana in Afghanistan: lo riconoscono i nostri alleati lo riconoscono i Ministri degli affari esteri e della difesa nel momento in cui convocano i vertici militari per ascoltarli sulle maggiori esigenze del nostro contingente militare. Ciò che abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedervi con insistenza è di mettere i nostri militari in grado di difendersi

di introdurre nel testo, ad opera di coloro che sono in grado di farlo, cioè il relatore o il Governo,

immediatamente ad eventuali motivate richieste dei nostri stati maggiori sull'adeguamento del contingente militare all'evoluzione della minaccia.

il motivo per cui non si voglia tener conto di una richiesta politicamente così impegnativa, a meno che non ci siano motivi ostatividi carattere politico che attengono esclusivamente agli equilibri interni della maggioranza.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo osservando, tuttavia, che gli articoli 1,

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti,

di emendamenti relativi all'incremento delle risorse affinché si possa svolgere quell'attività a favore delle comunità libanese, afgane e sudanesi.

La seconda ragione è che nelle nostre visite alle forze operanti in Libano e in Afghanistan abbiamo constatato come in realtà i risultati siano davvero pregevoli nello svolgere queste attività; la terza mira a raccogliere una voce diffusa e comune che vuole l'esaltazione dello sforzo italiano nel campo delle attività di sostegno allo sviluppo civile delle aree che sono in difficoltà. Debbo dire che, al di là di questa illustrazione, trovo - le sarei molto grato se mi ascoltasse un momento momento - veramente sorprendente che prima i relatori e successivamente anche il Governo abbiano avuto, secondo me, il coraggio di venire in Aula e di dire che siccome i tempi sono stretti non è il caso di emendare il provvedimento. Questa mi sembra una cosa che lei stesso non può accettare perché avalleremmo il discorso che il Senato rinuncia alla sua funzione legislativa peculiare perché è costretto da tempi ristretti, quando per ogni decreto, come lei bene sa, ci sono 60 giorni e quindi non potremmo spiegare a nessuno, al popolo italiano e a chiunque la ragione per la quale non debbano essere approvati degli emendamenti che consentano al Senato di svolgere la sua funzione legislativa.

Ministero degli esteri che da parte delle Forze armate per sostenere le popolazioni civili, fatto sbandierato e auspicato trasversalmente da tutte le parti politiche. Invito, quindi, ad una votazione responsabile.

Vede, Ministro, ieri il Presidente della Repubblica cui tutti ci richiamiamo ad ogni piè sospinto ha fatto appello alle intese tra i poli per quanto riguarda la politica estera. Credo che le intese - è questo il senso degli emendamenti che ho proposto all'Assemblea - riguardino anche le richieste che ogni parte propone all'Assemblea e la possibilità di vedersele approvate, perché altrimenti è un'intesa solo a senso unico.

lei al Senato ogni tanto viene e magari mette nei guai il Governo, com'è accaduto qualche settimana fa. Vorrei che oggi si evitasse tutto questo: questo: ieri ha detto che l'atteggiamento del centro-destra è vergognoso; oggi l'ha definito legittimo e questo lo considero un grande passo in avanti perché vuole dire che ha fatto un ragionamento e questa non è cosa di tutti i giorni. Noi abbiamo preparato alcuni emendamenti,

spero che su questo argomento la posizione di relatori e Governo rimanga quella che avevano manifestata in sede di Commissione. La questione riguarda innanzitutto non poche lire ma

la evidente ragione dettata dal calendario parlamentare che agli illustri colleghi non sfugge, essendo tutti esperti di lavori parlamentari. I colleghi, infatti, sanno bene che altro è il metodo adottato in prima lettura, altro è quello adottato in seconda. Al senatore Pisanu vorrei far osservare che una cosa è impegnare il Governo con un ordine del giorno a garantire l'idonea fornitura dei mezzi militari, altro è prevedere un simile impegno attraverso un emendamento. Si porrebbe quanto meno un problema di copertura che andrebbe

Si deve però far osservare che un conto è il finanziamento di prima istanza per far fronte all'emergenza, altro è il finanziamento in fase di *routine*.

Presidente, qui si pone un problema per quanto riguarda le risorse. Tutti, anche il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, sanno che il finanziamento previsto da questo decreto copre appena il 60 delle spese vive e non considera l'usura dei mezzi. Cosa significa questo? Significa che i mezzi che impegniamo ora in Afghanistan sono, non da mesi, ma da circa un anno usurati e devono essere o sostituiti o hanno bisogno di una radicale manutenzione. Poi dobbiamo anche ricordare, sempre per quanto riguarda le risorse finanziarie, che nell'ultima legge finanziaria sono stati tagliati ben 200 milioni di euro che erano diretti al finanziamento dell'addestramento delle nostre truppe e qui il Ministro della difesa dovrebbe anche dare qualche risposta al Parlamento. voglio ricordare anche ai pacifisti integrali che sono presenti in Aula che, in realtà, qui si sta svolgendo una commedia degli equivoci, signor Ministro, un pò come quella di quando il Presidente del Consiglio riteneva che la responsabilità delle decisioni sull'ampliamento della base della base di Vicenza ricadesse sul sindaco di Vicenza, oppure quando volevate far credere agli italiani che Karzai avesse deciso spontaneamente di liberare cinque talebani talebani perché era una sua decisione autonoma e non richiesta e sponsorizzata dal Governo italiano. Il problema è un altro e cioè che i pacifisti integrali, nel momento in cui hanno votato alcuni ordini del giorno, ed è giusto che questo il Paese lo sappia, hanno detto si all'invio di mortai da 120 millimetri, all'invio di elicotteri da combattimento Mangusta, ai blindati Centauro e Dardo e sostanzialmente a tutto quell'armamento di cui attualmente sono prive le nostre truppe, di questo si tratta. Quindi, bando alle ipocrisie, i pacifisti integrali in realtà, votando per quell'ordine del giorno e approvando l'adeguamento della presenza militare e della struttura militare, hanno votato anche per questo. Ed è giusto anche che qualche traccia rimanga nel corso di questo dibattito parlamentare.

*ad horas* cambia idea, da un momento all'altro, e quindi non possiamo fidarci.

ma questo spettacolo non infastidisce anche voi? Io credo di sì.

**Il Senato non approva.**

la lotta al narcotraffico e la distruzione delle coltivazioni e delle produzioni di oppio. Ciò serve ad affermare un punto decisivo della lotta contro il terrorismo di origine talebana.

anche se il provvedimento che uscirà difficilmente troverà d'accordo la Lega Nord, riteniamo quantomeno di limitare le perdite obbligando il Governo a riferirsi a degli organismi ben certificati e ben catalogati prima di disporre 40 miliardi di euro da spendere in modo del tutto arbitrario e discriminato.

la metà. Pertanto, a parte il rito burocratico che ha visto protagonista il relatore, per il fatto che non si possono disturbare i colleghi della Camera, vorremmo sapere se su tali questioni si può avere uno straccio di risposta politica.

Con l'emendamento 1.12, si propone di finalizzare la conferenza per i diritti umani delle donne e dei bambini a questioni di grande sostanza. L'85 per cento delle donne afgane

Presidente, anche questo emendamento corregge un'assegnazione veramente ridicola. Per un intero anno,

Avete svolto un'intera campagna per cinque anni, gridando alla differenza fra quanto speso per gli aiuti e quanto speso per le forze armate. Non riesco a capire per quale motivo dobbiate essere così bloccati.

Non si capisce perché, per tutte le iniziative delineate dall'articolo 1, il Ministro degli affari esteri non debba riferire in Parlamento come è invece previsto faccia per le iniziative

o ridurre qualche missione, chiedo che avvenga qui con una risoluzione, in chiave politica e non in chiave finanziaria. Questo è lo scopo per cui ho presentato questi due emendamenti. *(Applausi

in effetti, non ha torto nel sottolineare come il decreto preveda momenti di verifica e di informazione sulla parte militare e non sulla parte di cooperazione. Pertanto, propongo anche a lui, se intende, di trasformare l'emendamento 1.14 in un ordine del giorno. Il parere dei relatori è favorevole

Stiamo parlando, cioè, del sostegno e della cura a malati che sono orgogliosi di quello che ha fatto l'Italia per loro aprendo il Medical Centre di Baghdad. Mi consentirete in quest'Aula di rendere merito, per l'apertura di quell'ospedale, non al Governo di cui ho fatto parte, ma a un uomo coraggioso come Maurizio Scelli, che anche in quell'occasione rese onore alla nostra Patria. Signor Presidente,

la Camera dei deputati può bloccare l'approvazione del decreto, o lo approva in ventiquattro ore, visto che ha approvato un ordine del giorno, visto che anche la Camera è d'accordo? Perché, su un'azione di tipo umanitario si devono lesinare le risorse, che non vengono gestite da una ASL, ma della Croce rossa italiana? Chiedo all'Assemblea un attimo di raziocinio rispetto ad un emendamento del genere, di ragionare attorno ad un'operazione umanitaria, che serve a far sì che l'Italia possa vantarsi di una grande operazione di carattere sanitario e civile. SODANO non devi dirmi di calmarmi, perché è una vergogna che sia stata definanziata la Croce rossa per il mantenimento di questo ospedale. Questo ospedale davvero non è di destra o di sinistra, serve a curare i malati. Diamo, allora, al Senato la possibilità di chiedere alla Camera di approvare almeno una nostra modifica.

Signor Presidente, sappiamo che da più parti, anche autorevolissime, si insiste sulla necessità di rafforzare il nostro sistema di difesa in Afghanistan. L'emendamento che illustro è il 3.4, che si propone di mantenere la copertura finanziaria così come prevista, riducendo, però, il periodo da un anno, cioè «31 dicembre», a sei mesi, Il motivo di questa nostra proposta è finalizzato ad andare incontro alle esigenze di chi ritiene indispensabile rafforzare il nostro sistema di difesa. Si parla di *Predator*, sistemi assolutamente indispensabili di avvistamento elettronico, in grado di individuare qualsiasi nemico che possa operare sul territorio, di elicotteri Mangusta, anche questi assolutamente indispensabili. Si parla ancora, ministro Parisi, di rimettere in teatro gli AMX, inizialmente previsti. Si tratta di iniziative che servono per garantire la sicurezza del nostro contingente di terra in quello scenario. scenario. Proponiamo di modificare l'articolo 3, nel senso che ho anticipato, di ridurre cioè il periodo anziché ad un anno a sei mesi, come aveva sempre fatto il Governo Berlusconi nella precedente legislatura, andando incontro a quelle che allora erano le richieste di tutta l'opposizione, attuale maggioranza. Si chiedeva - e abbiamo sempre aderito - di ridurre, il periodo delle missioni a sei mesi. Con questo emendamento, riducendo il periodo a sei mesi ma mantenendo la stessa copertura finanziaria, di fatto la si raddoppia, andando incontro alle richieste di quanti chiedono maggiore aiuto finanziario per i nostri contingenti.

così da porla in condizione di creare disturbo una volta all'anno, anziché una volta ogni sei mesi. Questo è il motivo vero per cui ci viene proposta questa scansione temporale. Riteniamo assolutamente indispensabile tutelare la sicurezza dei nostri militari e il periodo di sei mesi è quindi anche finalizzato a consentire al Governo di mettere in atto tutte le iniziative anticipate dal ministro D'Alema per garantire la massima sicurezza al nostro contingente. del presidente Morando sull'emendamento 3.6. Presidente Morando, tutta Italia e chiunque stia assistendo a questo dibattito vede che l'opposizione fa delle proposte e voi le bocciate senza nemmeno discuterle, persino quando si tratta di malati. È un atteggiamento che Diliberto aggettiverebbe con termini a lui consoni. Io non mi permetto di dire qual è la sensazione che mi offre lo spettacolo della maggioranza che non vuole i voti del centro‑destra - questa è la realtà - e vorrei farlo notare al Capo dello Stato.

sia per quanto concerne l'autorizzazione alle spese delle missioni, sia per quanto riguarda l'impegno a riferire al Parlamento. Sul primo punto, osservo soltanto, per brevità, che se si anticipasse, come qui si propone, la cadenza (ora portata all'annualità) al semestre, si porrebbe il problema di rifinanziare nel secondo semestre le missioni qualora lo stanziamento si esaurisse nell'arco che va fino al 30 giugno. Sul secondo aspetto (cioè l'informativa al Parlamento), durante i lavori, soprattutto delle Commissioni, è emersa l'opportunità che le relazioni al Parlamento concernano, insieme, sia i risultati del mandato militare, sia i risultati del mandato civile

prevalga talmente sulle altre da oscurare l'importanza di missioni internazionali di grande rilievo, come ad esempio, quelle nei Balcani, di cui pochi si occupano in questo momento. Naturalmente, queste opportunità, che illustro nei termini più brevi data la mancanza di tempo, non richiedono una norma di legge, ma possono, se accettate dal Governo, orientare i nostri lavori per il futuro. gli emendamenti che ho citato il nostro parere è negativo, anche per le ragioni addotte dal senatore Tonini, che possono dispiacere perché in qualche modo limitano la deliberazione parlamentare ma che, se posso ricorrere ad una metafora letteraria, confermano l'insostenibile pesantezza dell'essere.

una temporizzazione semestrale per tutte le missioni. In particolare, sull'Afghanistan, dal momento che questo Governo propone al Parlamento l'indizione di una Conferenza di pace, presupponiamo che chi vuole la pace la voglia anche subito

contro. Ha già votato contro questo tipo di impostazione alla Camera e ha accettato l'allungamento al 31 dicembre, quindi, per coerenza di partito manteniamo questo atteggiamento.

Presidente, se ho capito bene, le parti separate riguardano la parola «Conseguentemente». Se salta il capoverso, ciò che segue non può più essere votato per parti separate.

Sono commi diversi e titolati a vivere per conto proprio, come prevede il Regolamento per le votazioni per parti separate. Peraltro, dello stesso parere

Signor Presidente, fornisco volentieri i chiarimenti che mi sono stati richiesti dal senatore Storace a proposito del parere formulato su questo emendamento dalla 5a Commissione permanente. L'emendamento 3.6 dispone una spesa palesemente priva di copertura finanziaria per il periodo successivo al 1° gennaio 2008. Il parere contrario è motivato molto facilmente con due argomenti: il primo è che l'espressione - ma questo sarebbe secondario - «in sede di manovra di bilancio» è completamente atecnica. Credo che si volesse dire «in sede di legge finanziaria per gli anni successivi». Se si sostituisse l'espressione "legge finanziaria" all'espressione che si usa nell'emendamento "manovra di bilancio",

È noto che nessuna legge ordinaria può stabilire quale debba essere il contenuto di una futura legge che il Parlamento approverà. Di conseguenza, nessuna norma che rechi un onere può essere coperta con riferimento ad una legge da approvare successivamente.

Potrei citare 100 precedenti che si trovano, presidente Morando, nel decreto Bersani. In Commissione affari costituzionali discutemmo sulla necessità ed urgenza di norme che rimandavano alla finanziaria; ne abbiamo viste di cotte e di crude. Sollevo però una questione politica,

In pratica, con l'emendamento che si propone all'Aula si dicono due cose: quando i Ministri vengono in Parlamento a riferire riguardo agli sviluppi delle operazioni militari e civili, si stabilisce che, ad esempio, riferiscano sulla destinazione dei fondi impegnati in attività di carattere non militare, cioè che fine fanno gli euro dati per le iniziative di carattere non militare. Ma la cosa più importante di questo emendamento, Presidente, è che esso impegna il Governo ad informare sulle valutazioni riguardo alla necessità di aumentare o meno i contingenti militari: cioè il testo di quell'ordine del giorno che vi è stato impedito di presentare, quello che riguarda la natura di ogni missione e la possibilità di decidere se vanno aumentati i contingenti militari o meno, diventa legge se approviamo questo emendamento.

Nessuno di noi, però, potrebbe mettere in discussione il fatto che servono delle protezioni personali adeguate solo per il semplice fatto che lì ti sparano addosso.

militare in tempo di pace, ma al codice penale militare di guerra, anche per consentire a questi ragazzi, che potrebbero sempre trovarsi sotto un fuoco di fila, di adottare almeno condotte conseguenti senza rischiare di veder

nel 1988 in occasione della missione della Marina militare nel Golfo Persico. Ricordo questo a puro titolo di vanità personale di cui faccio immediatamente ammenda.

L'inizio delle dichiarazioni di voto talvolta sembra essere la fine del secondo tempo di una partita,

l'Italia è da anni impegnata nelle missioni di pace: pace e guerra hanno ormai lo stesso significato. Guerre, con munizioni non convenzionali all'uranio impoverito: centinaia di migliaia di vittime civili e militari

hanno operato in quei luoghi con la stessa divisa che indossavano in Italia, a mani nude, respirando la terra sollevata dai carri armati. I militari americani e inglesi portavano tute speciali, maschere e guanti.

515 gravemente ammalati, alcuni terminali, di tumori, leucemie e quant'altro, signor Ministro, completamente abbandonati dal nostro Governo. C'è da non crederci: né cure, né pensioni, famiglie rovinate, madri impazzite. Un'altissima percentuale di militari al rientro dall'Afghanistan, è notizia di pochi giorni, dopo i risultati alterati delle analisi, sono stati operati alla tiroide per limitare i danni della contaminazione. Che futuro avranno? Questo cinismo, questo cinico disinteresse per la vita umana fa veramente paura. Oggi si chiede un «sì» al rifinanziamento delle missioni. Il no è chiaramente nella mia testa, nel mio sentire. Soldati, tutti a casa! Ma oggi ci troviamo con le bizzarre e contraddittorie astensioni di una parte dell'opposizione. In più, non posso dimenticare che ho preso un impegno con i molti che mi hanno votato: sostenere il Governo Prodi. Quindi, con non pochi problemi di coscienza, voto sì. Chiedo però che una legge europea condanni chi utilizza armi inquinanti a pagare i danni causati ai civili, ai militari e all'ambiente. Cindy Sheehan, la madre americana che ha perso un figlio in Iraq, è riuscita a mobilitare gran parte dell'America contro la guerra di Bush per il petrolio. Aspetto il giorno in cui tutte le donne del Parlamento italiano, in quanto donne e madri, si ribellino alla guerra che i governanti hanno nel loro DNA, votando un bel no alle cosiddette missioni di pace, una pace che per ora non ha portato né liberazione né democrazia ma solo miseria, dolore e morte.

Signor Presidente, come da tempo annunciato, voterò negativamente il decreto sulle missioni militari, il cui capitolo principale è il sostegno alla guerra in Afghanistan che, indipendentemente dalle furbizie parlamentari, trova, non a caso, il pieno sostegno delle destre che quella politica di guerra hanno avviato, politica di guerra e di distruzione. Ricordo che il presidente Bush parlò di ridurre quel Paese all'età della pietra, quel presidente Bush dal cui comando dipendono oggi le truppe della NATO e quindi anche quelle dell'Italia. Come è stato evidente, regole di ingaggio umanitarie differenziate da quelle americane in un teatro di guerra sono una contraddizione in termini: siamo in Afghanistan dentro il dispositivo militare della NATO per uccidere e per farsi uccidere. La situazione per il nostro Paese sta diventando sempre più compromessa: siamo percepiti come occupanti e l'*escalation* militare in corso rappresenta una via di non ritorno. Solo il ritiro del nostro contingente potrebbe far svolgere all'Italia un ruolo di pace e rendere credibile la proposta di una conferenza internazionale, altrimenti è pura ipocrisia e mera copertura della guerra. Ho votato contro tutti gli ordini del giorno della destra, che incrementavano la presenza bellica dell'Italia in quel Paese: la posizione che qui esprimo sul decreto è infatti la più lontana, abissalmente più lontana dalle forze della destra. Davanti alle nostre coscienze nessuna furbizia è possibile. In questo sono confortato dal pieno sostegno al mio voto parlamentare dell'associazione dei veterani di guerra americani del Vietnam e dell'Iraq, segno che la sensibilità per la pace sta crescendo anche negli Stati Uniti. In questo quadro, come già affermai un mese fa, confermo il mio appoggio esterno al Governo, ma confermo anche che di volta in volta deciderò le convergenze possibili. Da ultimo, il Governo italiano faccia ogni sforzo per restituire ai loro cari l'interprete di Mastrogiacomo e il mediatore di Emergency che ha consentito la liberazione del giornalista:

Dobbiamo uscire dal grande macello della guerra afghana. Ce lo impone la nostra Costituzione, ce lo chiede la grande maggioranza degli italiani e dovrebbe ancora guidarci (pur in tempi di cedimenti morali ed ideali verso la beatificazione del mercato e dell'affarismo) il DNA della sinistra e della cultura popolare (abbiamo fatto un indulto, che conteneva tanti elementi negativi, ma dicendo che ce l'aveva chiesto un grande tutti fingono di dimenticare che lo stesso Papa ci aveva anche chiesto di non fare la guerra). Quello afghano è un macello straziante e senza senso, in cui Berlusconi ci ha cacciato e da cui sbagliamo a non uscire. L'Afghanistan è il maggior produttore mondiale, oggi con noi che lo occupiamo, della droga, ne detiene il mercato e tutte quelle risorse vanno a finire dove vanno a finire anche i fondi della grande criminalità: nei paradisi fiscali. Ma oggi tra grande finanza e criminalità i confini sono sempre più labili.

e di come scavargli sotto ed a tale obiettivo purtroppo, oltre ai Casini *dona ferentes* lavora anche qualcuno del centro dell'Unione. Questa è la mia maggioranza, Prodi è il mio presidente del Consiglio, da cui vorrei vedere applicato tutto il programma elettorale e non solo le parti peggiori di quel compromesso. Così come avrei voluto, insieme a tanti salariati, impiegati, precari e pensionati italiani, che avessimo questa volta evitato, come troppe volte è successo,

e dai venti di guerra che spirano sull'Iran. L'unico modo di salvare i nostri soldati è portarli a casa.

responsabilità, dignità e credibilità sono le tre parole chiave che sintetizzano efficacemente le ragioni del sì convinto dell'UDEUR alla legge di conversione del decreto n. 4 del 2007. Tale decreto assicurerà, per l'anno in corso, la prosecuzione degli interventi e delle attività destinate a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, prevedendo altresì la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle forze di polizia alle numerose missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario vedono impegnato il nostro Paese. Responsabilità, dignità e credibilità perché l'Italia ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione di alcuni conflitti internazionali cui non può assolutamente venir meno, perché la classe politica su questioni quali quelle di politica estera ha il dovere di superare diatribe di partito o di schieramento e di tentare di esprimersi in maniera chiara e univoca in nome dei valori della patria, che sono ben al di sopra delle sterili contrapposizioni di parte. Ritengo dunque incomprensibile l'atteggiamento dell'opposizione, non solo riguardo al decreto, sul quale ha deciso di astenersi, ma anche sulla vicenda Mastrogiacomo, anche perché il Governo oggi ha dimostrato ampiamente la volontà di instaurare un dialogo sereno e non strumentale su questioni delicate e di voler chiaramente assumere responsabilità e impegni seri per garantire la sicurezza del personale civile e militare in Afghanistan,

probabilmente nel modo più sbagliato possibile, assoggettando la decisione a mere logiche di politica interna, quando fino a dieci giorni fa il percorso su questo decreto di rifinanziamento era normale. una missione che non nasce con questo Governo e con questa maggioranza, è una missione che nasce con il precedente Governo. Ce lo avete insegnato voi, amici della Casa delle Libertà: in politica estera ci si impegna a nome di tutta la Nazione. E noi ci siamo fatti carico di andare avanti in questa missione che ci veniva chiesta dall'ONU, dalla comunità internazionale e dalla giovane democrazia afghana. Fino a qualche giorno fa era tutto normale, poi non si è capito più cosa sia successo, quasi come se una decisione così impegnativa in politica estera, che fa riferimento alla credibilità che la nostra Nazione ha nel rapporto con le altre Nazioni, a un certo punto sia diventata oggetto di politica nazionale, e quindi si è intravista ancora una volta la sempre solita storia del tentativo di dare la spallata. Ritengo che facciamo un torto ai nostri ragazzi

far prevalere l'interesse collettivo rispetto all'interesse di parte. Non sempre ciò è facile. Noi abbiamo difficoltà su questi provvedimenti eppure riusciamo a governare al nostro interno, ma è chiaro che nel momento in cui vengono difficoltà poste da un'altra parte probabilmente si gioca ad accentuare le nostre difficoltà. Questo non è giusto e soprattutto credo non sia giusto in politica estera. Concludo, Presidente, confermando il voto favorevole dei senatori e delle senatrici dell'Italia dei Valori ad un provvedimento che ci viene chiesto dalla comunità internazionale e dall'ONU, ma soprattutto ad un provvedimento che mantiene il livello della credibilità esterna dell'Italia

Presidente, in sede di dichiarazione di voto, nella fase conclusiva cioè del dibattito sul decreto di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali, pur essendo pur essendo ed essendo stati favorevoli a dette missioni, non crediamo si possa dare una valutazione del decreto stesso prescindendo dal considerare i fatti verificatisi negli ultimi giorni sul fronte più caldo in cui opera una delle nostre missioni, quello afghano, e sugli atteggiamenti in proposito assunti dal Governo, con le conseguenti ripercussioni sui nostri rapporti con i Paesi alleati. Due domeniche fa, mentre era in corso il sequestro del giornalista de «la Repubblica», un acuto osservatore politico, non certo classificabile come portavoce berlusconiano, Angelo Panebianco, scriveva: «La coincidenza tra l'offensiva alleata nel Sud dell'Afghanistan e il sequestro dell'inviato de "la Repubblica", Daniele Mastrogiacomo, sta cambiando il significato della nostra presenza militare in quel contesto. La situazione è precipitata e quella che ancora poche settimane fa si poteva presentare come una missione di pace e di ricostruzione dell'Afghanistan si mostra per ciò che di fatto è o è diventata, una missione di guerra, benedetta dall'ONU a fianco dei nostri alleati occidentali. Nel dibattito italiano» - proseguiva Panebianco - «le vere poste in gioco vengono raramente menzionate. La prima riguarda il duello tra Occidente e terrorismo islamico. Se i talebani riprenderanno il controllo dell'Afghanistan, la galassia terroristica avrà conseguito una vittoria straordinaria (...). La seconda posta in gioco riguarda la sopravvivenza della NATO.

DEL PENNINO). Ma il richiamo alla gravità della situazione e all'esigenza di un più forte impegno sul fronte afghano lo troviamo anche nella bella relazione con cui il collega Tonini ha illustrato il disegno di legge di conversione del decreto alla nostra Assemblea, anche se le sue considerazioni sono volte a enfatizzare il ruolo dell'eventuale conferenza di pace. Dice, infatti, il senatore Tonini che la situazione afghana presenta numerosi elementi di preoccupazione: tutti gli osservatori convengono nel registrare una tendenza al peggioramento e si è aperta, di conseguenza, una discussione sulla necessità di rafforzare l'impegno militare della NATO e di rivedere le regole d'ingaggio

che in Afghanistan, all'inizio dell'inverno, c'erano schierati dalla NATO, su mandato ONU, in tutto 36.000 uomini, uno ogni 25

40.000 uomini, uno ogni 0,3 chilometri e ogni 50 abitanti. Egli ha concluso che per questo motivo l'invio di maggiori truppe e di più forti interventi è assolutamente indispensabile. Rispetto a queste oggettive considerazioni e a questa oggettiva analisi della situazione, qual è stata la linea del Governo e della maggioranza? Potremmo definirla la linea di Chamberlain. Ha cominciato l'onorevole Fassino, che è vero che non fa parte del Governo, ma è pur sempre il segretario del maggior partito della coalizione, che ne rappresenta fra l'altro l'ala riformista e che si può dire sia anche l'interfaccia partitico del Ministro degli affari esteri, il quale Fassino ha proposto di far partecipare i talebani alla futura ipotetica conferenza di pace. Ora, l'intervento in Afghanistan, come ricordato nella sua relazione anche dal senatore Zanone, fu deciso all'indomani dell'11 settembre dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con la risoluzione 1368 per sottoporre a giudizio autori, organizzatori e sostenitori di attacchi terroristici, associando alla responsabilità quanti offrissero loro sostegno ed aiuto. I talebani erano, e sono, sostenitori degli attacchi terroristici e hanno dato rifugio ai loro esecutori. Nulla quindi di più improvvido che proporre di fare dei talebani interlocutori di un processo di pace, riconoscendo loro la qualifica di legittimi combattenti. Non sappiamo se ha fondamento il dubbio, sollevato da un altro commentatore politico, che la proposta di Fassino rappresentasse un messaggio ai talebani per favorire la liberazione di Daniele Mastrogiacomo. L'errore politico di quella proposta rimarrebbe intatto, anche se nobilitato, ma per certi versi aggravato dall'intento umanitario. Che l'estemporanea uscita dell'onorevole Fassino non rappresentasse soltanto un incidente di percorso di questa maggioranza è confermato dal successivo atteggiamento del Governo italiano nelle trattative sul sequestro Mastrogiacomo.

Questa scelta ha inevitabilmente comportato un esito che ha determinato un cedimento rispetto ai tagliatori di gole talebani, del quale non è difficile prevedere le ulteriori conseguenze. Non a caso, le reazioni di tutti i Paesi alleati sono state pesantemente negative. Non mi riferisco tanto alle posizioni assunte dal Dipartimento di Stato, rispetto alle quali è facile l'obiezione della sinistra antagonista, e non solo, che rivendica l'autonomia che rivendica l'autonomia dell'Italia in una logica europea rispetto all'egemonismo americano. Piuttosto, mi riferisco alle prese di posizione proprie degli alleati europei. Il portavoce del *Foreign Office*,

onorevole Bonino ha esplicitamente dichiarato che la «reazione pubblica degli Stati Uniti è comprensibile. La liberazione di cinque talebani, che le truppe NATO rischiano di trovarsi di fronte nei ranghi dei nemici armati, è questione della quale vanno valutate le conseguenze».

Alla luce di queste oggettive considerazioni, appare del tutto evidente che non è possibile considerare frutto di un pregiudizio dei Gruppi dell'opposizione l'affermazione che siamo in presenza di una politica estera equivoca e contraddittoria da parte del Governo. Questo carattere equivoco e contraddittorio della nostra politica estera è confermato dall'iniziativa del sottosegretario agli Esteri Vittorio Craxi che, in violazione dei principi fissati dal Quartetto e dall'Unione Europea, si è premurato di assicurare al Primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese, esponente di Hamas, l'impegno dell'Italia ad appoggiare lo stop all'embargo, e questo senza essere smentito né dal Presidente del Consiglio né dal ministro D'Alema. La verità è che il Governo, stretto fra la conclamata fedeltà all'alleanza internazionale del Paese richiesta dalla sua componente riformista e le spinte antiamericane e di pacifismo militante interpretate dalla sinistra antagonista che ne è parte essenziale, non è in grado di garantire una coerente linea di politica estera. Oggi, non è nemmeno in grado di garantire l'unità della sua maggioranza sulle proprie contraddittorie scelte internazionali. Non a caso, mentre nel luglio scorso, in occasione del voto per il rinnovo delle missioni internazionali, respinse sdegnosamente i voti dell'opposizione e ricorse alla fiducia, oggi, sapendo che nemmeno apponendo la fiducia su questo provvedimento potrebbe garantirsi un'autonoma maggioranza, invoca il sostegno delle opposizioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto tengo a esprimere personalmente tutta la mia gioia e il profondo sollievo per l'avvenuta liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo. Ringrazio sia il Governo, sia l'associazione umanitaria Emergency. Al tempo stesso, tengo a esprimere il nostro cordoglio alla famiglia del giovane autista afgano che, purtroppo, è stato barbaramente ucciso. Oggi quest'Aula è chiamata a votare sul decreto che rinnova i finanziamenti per le missioni internazionali all'estero, dunque anche quella che riguarda la controversa missione italiana in Afghanistan. A tale riguardo, intendo ribadire che il Gruppo per le Autonomie si è sempre e fermamente dichiarato contrario all'uso della forza per la risoluzione dei conflitti. Le guerre non solo non contribuiscono in alcun modo alla pacificazione e stabilizzazione delle zone di conflitto, ma sono fortemente dannose; basti pensare all'attuale *escalation* di violenza in Iraq. Anche chi era a favore, a suo tempo, adesso deve ammettere che si è generato un disastro con l'attacco militare degli Stati Uniti appoggiato da parecchi Stati europei. Soprattutto nelle province meridionali e orientali dell'Afghanistan, la pressione militare dei talebani è infatti in netta ripresa. Prova ne è che la forza internazionale ISAF, sotto comando NATO, è passata da 9.000 a 31.000 uomini circa. Con l'intento di anticipare la preannunciata offensiva di primavera dei talebani, la NATO ha dato inizio, lo scorso 6 marzo, alla più massiccia operazione militare (l'operazione Achille) in terra afgana dal 2001. Signor Presidente, ne siamo consapevoli tutti: lo scontro sta diventando sempre più feroce e si sta estendendo anche a quelle province ritenute fino a qualche mese fa «tranquille», come Herat, dove è situata la base occidentale del contingente italiano. Il rischio di attentati continua a essere molto elevato. Nelle prossime settimane sarà guerra a tutto campo, specialmente nel tormentato Afghanistan del sud. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna chiedono agli alleati della NATO di aumentare il proprio contingente. Reagire al divampare di questo scontro con una risposta militare ancora più dura sarebbe, tuttavia, un tragico errore che non solo non risolverebbe nulla, ma sarebbe controproducente e causerebbe sempre più vittime. Tengo a ricordare che il conflitto in Afghanistan ha già ucciso un paio di migliaia di persone. Secondo lo *Human Rights Watch* oltre mille civili sono morti nel solo 2006 per gli effetti collaterali della guerra tra le forze ISAF e i talebani. E la morte di questi civili non fa altro che fornire un'ulteriore base di odio alle tensioni già esistenti. Questa *escalation* di violenza ci obbliga, pertanto, a investire in un cambio radicale di strategia. Dobbiamo imprimere una svolta in questa terra martoriata da anni dalla guerra. Deve finalmente cambiare l'intervento diplomatico. Dobbiamo aumentare la cooperazione civile e le risorse, affinché l'Afghanistan possa affrontare le grandi difficoltà economiche e sociali. Soltanto in questo modo si può arrivare a una stabilizzazione politica duratura. Prendiamo atto con soddisfazione che il Governo italiano si è detto fin da subito contrario a un impegno maggiore di truppe. Il ministro degli affari esteri Massimo D'Alema ha confermato la scorsa settimana in sede ONU che la presenza militare italiana resta limitata limitata alle province del Nord-Ovest e che 2.000 soldati è il massimo che il nostro Governo possa permettersi. Come ho già detto, per superare la crisi afghana dobbiamo trovare vie alternative alla guerra. Siamo fieri che l'Italia, tramite il nostro Governo, si sia fatta promotrice di una Conferenza internazionale di pace. Ringraziamo il ministro degli affari esteri D'Alema e tutto il Governo per averla richiesta con fermezza al Consiglio di sicurezza. Essa è l'unica realistica strada per tentare di stabilizzare e pacificare questo tormentato Paese. Per riuscire in questo intento, tuttavia, è necessario coinvolgere tutte le parti in causa, disposte, naturalmente, a collaborare per trovare una soluzione duratura e pacifica al conflitto afghano. Soltanto un confronto leale con tutte le parti interessante, che non deve escludere la durezza, può, a nostro avviso, fornire uno spiraglio per la democratizzazione del Paese. Per concludere, signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al disegno di legge in esame, perché il multilateralismo è al centro della politica estera di questo Esecutivo, ma soprattutto perché esso si è fatto promotore di una conferenza internazionale di pace. Infatti, il decreto legge autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 per l'organizzazione nell'ambito delle Nazioni Unite della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal nostro Esecutivo. Inoltre il provvedimento prevede un aumento di risorse finanziarie da destinare in aiuti umanitari. Degna di nota è soprattutto l'autorizzazione di spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini nei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto-legge. Al tempo stesso ribadisco, però, la necessità di una politica estera, la quale deve prioritariamente valorizzare gli strumenti di prevenzione dei conflitti, di mediazione e di accompagnamento dei processi di pace.

e per un suo protagonismo sulla scena internazionale. Il nostro Paese deve far sì che l'Unione europea sia forza di pace, di libertà, di democrazia e di sviluppo per far rispettare la legalità ed il diritto internazionale. *(Applausi dai Gruppi Aut

Osama Bin Laden e gli altri di Al Qaeda sono liberi e seminano terrore. Hanno rafforzato il loro potere non solo in termini militari, ma - ed è questa, a nostro parere, la sconfitta più grande anche diventati un punto di riferimento per tanti afghani e da molti vengono visti come coloro che si battono per la liberazione del Paese. Il terrorismo è aumentato, l'azione dei kamikaze è arrivata fin lì. Io la vedo come una sconfitta. Per chi, come noi, non ama gli integralismi - neanche quelli di casa nostra, per capirci - e si batte per la libera scelta di ogni individuo, a qualsiasi sesso, razza, religione appartenga, i talebani rappresentano l'oscurità, la negazione della vita. Siamo sgomenti nel vederli più forti e più minacciosi. Ma anche i signori della guerra sono diventati più forti. Il commercio dell'oppio, come è stato detto da tantissimi, non è mai stato così imponente. Se la situazione è questa, tutti - anche l'opposizione - dovrebbero capire che non esiste una possibilità di soluzione militare. Tutti dovrebbero ragionare seriamente senza strumentalismi, che invece abbondano in maniera anche micidiale in alcuni momenti,

a tentare altre strade, si batta per la Conferenza internazionale di pace. E quella Conferenza, difficile, tutta ancora in salita, viene attaccata e interpretata da alcuni come un patetico tentativo di tenere a bada la cosiddetta sinistra radicale. La verità è un'altra: la Conferenza internazionale di pace è una proposta di grande valore e io sono grata al Governo e al Ministro degli affari esteri per essersi battuti. È però una proposta che incontra consensi, ma anche molte diffidenze e ostruzionismi. vengono soprattutto da chi ha investito nella guerra come strumento capace di risolvere ogni conflitto. Solo che la guerra con costruisce nessuna relazione: semina odio, rancore, divisioni. Il mondo è diviso da assurde guerre di civiltà che si fanno strada con la prevaricazione, l'occupazione, il bombardamento di popoli inermi e innocenti. Qualcuno, anche tra i più accaniti tifosi di Bush (ce ne sono in Italia e anche in quest'Aula), potrebbe dire che dire che la guerra in Afghanistan ha dato risultati? Che a distanza di sei anni non si è ulteriormente inasprita? È una guerra sbagliata, nei fatti persa. È una drammatica testimonianza, assieme all'Iraq, dei guasti provocati dalla guerra preventiva. Noi non ci rassegniamo, ci consideriamo cittadini di un Paese autonomo, che ha la sua politica e fa le sue scelte. Per questo apprezziamo gli atti del Governo e, nella misura in cui possiamo, lo stimoliamo. Vediamo bene quanta distanza c'è tra la politica estera del Governo Prodi e quella del Governo Berlusconi. Ci hanno molto turbato, onorevoli senatori, le strumentalizzazioni sul caso Mastrogiacomo e sul tardivo (diciamo così) dissenso degli USA rispetto alla trattativa. Gli USA hanno trattato per gli americani prigionieri, hanno scambiato prigionieri, hanno dato soldi e hanno fatto bene se questo è servito a salvare delle vite umane. In quest'Aula si fa tanto spesso appello alla vita umana, alla sua sacralità, alla sua intoccabilità. Perché due pesi e due misure? Perché una tale asimmetria di valori? Si grida allo scandalo alla sola idea della presenza dei talebani alla conferenza internazionale quando persino il Ministro degli esteri di Karzai non chiude a questa prospettiva, pur ponendo, giustamente, delle condizioni. Ma i talebani non sono stati nel passato uno strumento degli USA? Non sono stati foraggiati e addestrati? E oggi lo sono anche dal Pakistan, dove c'è un Governo amico degli americani. Credete davvero che Karzai avrebbe fatto una trattativa tenendo all'oscuro gli Stati Uniti d'America? Noi - Verdi e Comunisti italiani - abbiamo infiniti problemi a votare il rifinanziamento della guerra in Afghanistan, ma vediamo i passi avanti, incerti, difficili, anche complicati, che si stanno facendo e, sconcertati, ma come può, chi crede alla dignità nazionale, volere un Governo trattato come un suddito che deve obbedire tacendo, addirittura rafforzando il proprio impegno in una guerra fallita? Leggo un po' così, in parte, gli ordini del giorno per i nuovi armamenti che, in qualche modo, sottintendono anche nuove regole di ingaggio. A noi sta a cuore la vita dei nostri soldati, molto, tantissimo, come ci stanno a cuore tutte le vite. Il Governo valuterà, assieme ai militari impegnati, se rafforzarne la difesa. Ma voi chiamate le cose con il loro nome. Quando chiedete più armi voi, in realtà, pensate ad un ruolo diverso dell'Italia in Afghanistan: un ruolo attivo, di guerra, di bombardamenti, non ai talebani, che se ne stanno ben rinserrati su montagne irraggiungibili, ma su civili inermi, su un Paese ormai stremato dalla povertà. Noi abbiamo a cuore - lo ripeto - la vita delle persone e votiamo a favore perché vogliamo accompagnare gli sforzi del Governo per la Conferenza internazionale di pace e perché abbiamo apprezzato moltissimo quanto fatto per la liberazione del giornalista de «la Repubblica». Saremo al fianco del Governo perché la Conferenza di pace si faccia e rappresenti una tappa contro una guerra in cui si bombardano villaggi costruiti con il fango.

mi ascoltasse, mi farebbe un favore. Dicevo che chiediamo un'iniziativa forte che, al di là delle strumentalizzazioni e del fango gettato su un'organizzazione come Emergency, dia il segno di come intendiamo la vita, la riconoscenza, se mi è permesso usare questo termine. Due uomini, l'interprete di Mastrogiacomo ed il mediatore di Emergency, rischiano di essere uccisi. Hanno messo in gioco la loro vita in due missioni: uno per aiutare Mastrogiacomo a raccontare cosa succede quando le bombe hanno la meglio sulla ragione; l'altro, per aiutare il nostro Paese nella liberazione di Mastrogiacomo. Signori del Governo, meritano di essere salvati, dovete riuscirci e noi vi affiancheremo con lealtà e solidarietà. Lo dobbiamo a quei due uomini. È il Paese che glielo deve.

che non ci convincono, che non ci hanno convinti, anche nelle dichiarazioni del Ministro degli affari esteri. Innanzitutto, colleghi, è accaduta una cosa stranissima. Noi pensavamo di sapere cosa fosse la fiducia, però ci siamo sbagliati: non esiste solo la fiducia che pone un Governo per tagliare la discussione e non consentire nessuna interferenza parlamentare sui propri provvedimenti. Abbiamo visto che esiste anche anche un'impropria fiducia quando non c'è tempo. Il Governo avanza la questione: non abbiamo tempo per discutere, per emendare, *ergo* si respinge tutto, anche ciò che si dice essere opportuno, giusto e condiviso. È una cosa aberrante, lo hanno già detto alcuni colleghi, davvero impensabile. Non ci convincono tanti discorsi che abbiamo sentito. La metà dei partiti della sinistra italiana da anni continua a dire: tutti a casa i militari, tutti a casa i militari (questo era il loro motto) nelle piazze piene di bandiere colorate. Oggi dicono, con un ragionamento astruso, con una premessa negativa, che dovranno votare il provvedimento per responsabilità nei confronti di un Governo che sembra abbia fatto chissà cosa di nuovo in politica estera se non perpetrare esattamente quello che era stato fatto dal Governo precedente. L'unica persona onesta, probabilmente, che si è autoconfessata, è stata il collega Turigliatto che ha detto: è inutile giocare con le furbizie, diciamo come stanno le cose, nel senso che o le condividiamo o non le condividiamo; ma non possiamo dire che non le condividiamo però *obtorto* *collo* le dobbiamo votare perché nessuno qua vuole andarsene a casa, perché se cade un'altra volta un Governo sulla politica estera, non c'è unità del Paese, non c'è una maggioranza sulla politica estera, è giusto andarsene tutti a casa. Ma è quello che chiede il Paese, sapete? È quello che chiedono per tutte le strade i nostri elettori. Non ci piace nemmeno (qui c'è un collega quasi di casa ne ha appena parlato, il senatore Peterlini) questo avere eletto ad eroe un giornalista liberato. Premesso che tutti siamo felici tutti siamo felici - perché la sua famiglia ha potuto riavere i propri affetti. Cari signori, cito il collega Peterlini perché abitiamo nelle stesse zone montane e pur conoscendo noi cosa è la solidarietà alpina quando uno scellerato alpinista - ripeto, uno scellerato alpinista - improvvidamente, per propria imprudenza, si espone a rischi esagerati

A noi viene chiesto un voto su questo provvedimento di rifinanziamento delle missioni militari italiane all'estero, che però sottende due domande, purtroppo, e noi dobbiamo dare una sola risposta. La prima domanda è se è giusto che i nostri militari siano impegnati su un territorio dove si addestrano e si organizzano i terroristi, che colpiscono tutto l'Occidente. Si tratta di nemici che in questo momento controlliamo,

Riassumendo la nostra posizione, sottolineo che non siamo soddisfatti del dibattito, dell'informazione, delle intenzioni poco chiare

L'UDC si tiene coerente alla linea che ha sostenuto fin dal mese di agosto dello scorso anno quando, superando ogni esitazione e remora determinate da posizioni intestine all'attuale maggioranza, ha innanzi tutto ritenuto, non per rendere un servizio al Governo e alla maggioranza (perchéquesto non ha fatto,

La politica estera, pur libera dai vincoli che l'Italia ha conosciuto e ha sopportato negli ultimi 50 anni, proprio perché più libera può scegliere di onorare le proprie alleanze, di rimanere coerente, seria e leale rispetto agli impegni assunti in sede internazionale, può in buona sostanza porsi come la piattaforma di convergenza del popolo e dell'intera Nazione, prima ancora che delle forze politiche. Si usa dire che la politica estera debba essere *bipartisan*. Questo per noi è un valore; lo è a maggior ragione nel momento in cui l'Italia è impegnata in più missioni. Il dibattito che si è svolto in Senato é stato risucchiato prevalentemente dal tema Afghanistan, eppure sarebbe stata necessaria una qualche considerazione su missioni nelle quali siamo impegnati nei Balcani o in Libano, entrambe delicatissime, o su altre situazioni che si prospettano

Qui è giusto ricordare che è nella tradizione della democrazia italiana e della democrazia repubblicana un internazionalismo democratico - uso questo termine che evoca altri internazionalismi, ma se ne differenzia proprio per le ragioni della pace, al punto che tutte le missioni italiane sono state missioni di pace. Per tornare all'Afghanistan, una missione in questo territorio è senz'altro di pace, ma non può essere una missione disarmata. Ora, dall'approvazione del decreto‑legge alla Camera ad oggi sono intervenute alcune vicende sulle quali dovrò necessariamente soffermarmi sia pure brevemente. Alla Camera soltanto i colleghi della Lega hanno tenuto una posizione diversa all'interno dello schieramento delle opposizioni, perché è inutile dire che ci sono più opposizioni. La Lega alla Camera si è astenuta. Oggi - a me e a noi rincresce - altre forze d'opposizione scelgono questa linea della astensione. Per noi, invece, sarebbe stato giusto mantenere, nonostante le vicende alle quali adesso mi richiamerò, costante e coerente la linea del voto favorevole al provvedimento che finanzia la missione separando in ogni ragionamento sulla politica estera, che dovrà trovare in un momento successivo all'attuale anche occasioni di verifica e di approfondimento, l'impegno

che all'interno della maggioranza - ne é stata profonda testimonianza il discorso che abbiamo ascoltato poc'anzi dalla senatrice Palermi - esistono non delle sfumature, ma delle grandi differenze di valutazione delle grandi differenze di valutazione per le quali la presenza in Afghanistan non è voluta allo stesso modo con cui è sostenuta dal Governo o, meglio, dal Ministro degli esteri e dal Ministro della difesa che hanno una responsabilità istituzionale. Non ci siamo lasciati prendere e non ci lasciamo prendere da queste differenze. Riteniamo che il provvedimento vada egualmente votato e tuttavia non possiamo fare a meno di precisare che quanto è avvenuto dal voto della Camera ad oggi ha una nostra precisa valutazione politica. Che cosa è avvenuto? Innanzitutto, il sequestro e la liberazione di Mastrogiacomo. Abbiamo chiesto, sin dal primo momento - lo ha fatto il presidente del nostro partito onorevole Casini - che il Governo si adoperasse e si impegnasse per la liberazione di Mastrogiacomo.

che per non pochi (certamente per molti che siamo stati democristiani o lo siamo rimasti nell'animo) la disponibilità ad aprire anziché il fronte della non trattativa quello della trattativa non ha rappresentato una scelta facile.

sui quali una valutazione più compiuta e più approfondita andrà svolta nel corso del tempo, senza interferire nella discussione e nella votazione che dovremo affrontare oggi. oggi. Ci sono, infatti, effetti collaterali che richiamano certamente e pongono l'esigenza di una precisazione del senso della nostra presenza in Afghanistan. È una missione di pace, ma non può essere una missione disarmata sino al punto di subire il primo, il secondo ed il terzo attacco. Non può essere una missione disarmata cui non si interviene nel caso in cui ci sia una offensiva dei talebani. E può anche venire il dubbio che il primo episodio di tale offensiva sia stato rappresentato anche dal sequestro Mastrogiacomo

La mozione dell'ONU con cui si impegnano i Paesi che poi hanno scelto di recarsi in Afghanistan vincola alla difesa del Governo Karzai. Senza la difesa di questo Governo viene meno un elemento della missione di pace: la ricostruzione dell'equilibrio politico, difficilissimo per le circostanze per le quali l'Afghanistan è tra è tra l'Iran e il Pakistan, Paesi che hanno storicamente interessi che si sono sempre espressi nella direzione della egemonizzazione, per non dire della conquista, del Paese. Orbene, noi sappiamo che i talebani non sono un nostro nemico; sono un nemico dell'Afghanistan. Se vogliamo un Afghanistan libero e democratico, con quella democrazia che tutti abbiamo apprezzato quando larga parte del popolo afgano è andato a votare, dobbiamo riconoscere che è su questa linea che dobbiamo rimanere seri ed impegnati. In conclusione, non posso non rivolgere un appello anche alle altre forze dell'opposizione. Si tratta di una scelta pregiudiziale con obiettivi politici di carattere diverso, rispettabili. Anche noi vogliamo presto la crisi di governo, ma non possiamo determinare una difficoltà delle missioni oggi. E noi facciamo nostra, onorevoli colleghi - lo voglio ricordare - l'affermazione dell'onorevole Berlusconi al momento del voto della missione in Kosovo, quale così si espresse: «La nostra coscienza ci impone di mettere il nostro Paese in condizione di rispettare gli obblighi liberamente assunti, di tener fede all'alleanza e di onorare i trattati sottoscritti. È il sostegno che ancora una volta siamo pronti a dare all'Italia nel pieno esercizio della nostra responsabilità e nella consapevolezza dei doveri che spettano anche all'opposizione

Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, annuncio, a nome di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, il voto a favore della conversione in legge di questo decreto.

e molto importante dell'Unione e per volontà del popolo, come seconda componente dell'Unione stessa, per cui siamo un Gruppo di un qualche interesse, di una qualche importanza. Veniamo definiti in vari modi, più o meno pittoreschi, ma quello che ci caratterizza è che abbiamo scelto questa posizione e che il popolo ha confermato per noi un significativo ruolo in questa posizione. Tuttavia, il nostro voto non è tranquillo, è un voto insieme ragionato e critico, preoccupato e responsabile, anche sofferto. Penso che non potrebbe essere diversamente: la situazione è talmente complicata, drammatica e difficile che soltanto una leggerezza veramente incomprensibile o la piccineria di appassionarsi prevalentemente a piccoli giochi di potere, potrebbe far votare un argomento di questo genere a cuor leggero. Mi Mi tratterrò brevemente su due soli punti, potendo tener conto naturalmente degli importanti interventi che nel corso del dibattito altri colleghi di Rifondazione hanno reso in quest'Aula: prevalentemente il caso Mastrogiacomo e, naturalmente, l'Afghanistan. Devo dire che sul caso Mastrogiacomo, più ancora di quanto il senatore Tonini ha detto oggi, per noi rimane assolutamente approvabile in tutto e per tutto quanto egli disse una decina di giorni fa, proprio quando se ne parlò in

su tutto tranne ciò che non è negoziabile, e non lo è la caratteristica della missione e la sua finalità. Questo mi pare assolutamente accettabile, molto importante. Dirò rapidamente: Tonini *locuto*, causa finita per noi, siamo del tutto d'accordo. Ma cosa significa questo? Significa, per l'appunto, che rivendichiamo anche una caratteristica della nostra tradizione nazionale e popolare che è quella di distinguere attentamente, di volta in volta, fino a che punto ci si può spingere. È stato citato spesso il caso Moro: io me lo ricordo bene, tra l'altro con Rina Gagliardi, Rossana Rossanda e altri noi eravamo per la trattativa, come i socialisti, come Sofri, come più di uno, e mi ricordo di avere allora scritto su "il manifesto" che i Nazisti trattavano con noi: ci chiamavano banditi, ci sparavano a vista senza processo se sforavamo di 20 minuti il coprifuoco, ma quando noi catturavamo un soldato della Wehrmacht trattavano con noi perché pensavano che fosse in gioco qualcosa di particolarmente importante persino per loro. Nella città dove io ho lottato nella resistenza, Novara, per noi trattava il vostro vescovo, monsignor Orsola, un famoso vescovo, e trattava a dimostrazione del fatto che queste cose sono sempre piene di ambiguità e di ritorni all'indietro: i nazifascisti misero un milione di taglie sulla sua barba, era un frate cappuccino, e gli bruciarono l'automobile. Allora io penso che ogni qual volta ci troviamo in queste vicende, dobbiamo saper sempre tenere conto che ci sono alcuni punti non negoziabili e per tutto il resto bisogna avere il massimo di abilità e anche di scaltrezza e anche persino di incapacità di tener conto di scrupoli perché questo è assolutamente necessario. A questo punto siamo contenti, molto contenti e contente che Mastrogiacomo sia libero. Non capisco per quale ragione, repentinamente, chiunque altro si trovi in difficoltà è scomparso dalla scena: per esempio il rappresentante di Emergency che ancora si trova prigioniero sembra che non interessi più a nessuno. Noi invece aggiungiamo il nostro appello a quello che viene fatto da Gino Strada e da altri perché anche di lui ci si occupi. occupi. Questo è il punto per quello che riguarda Mastrogiacomo. Appartiene alla nostra sovranità nazionale, che è un aspetto della nostra sovranità popolare, anche avere caratteristiche specifiche nel trattare questi argomenti: i tedeschi trattano di meno, i francesi trattano abbastanza. Dipende sia dalle circostanze, che dalle tradizioni popolari. L'importante è che non venga messa in dubbio la finalità della missione. Per questo già in quel che ha detto il senatore Tonini era presente la posizione del Governo, che mantiene ferma la missione. Sono convinta, oltretutto, che persino spingerla, per motivazioni anche giustificate o comprensibili, verso altri lidi, ossia un aumento della sua caratteristica militare, sarebbe anche incostituzionale, perché dell'articolo 11 non c'è soltanto il secondo comma, c'è anche il primo, che afferma che ripudiamo la guerra non solo come offensiva, ma anche come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Dunque, la nostra Costituzione ci fa obbligo di cercare altri strumenti di risoluzione delle controversie internazionali, sempre e in ogni momento: appena si apre una crepa, una possibilità, una incertezza, una difficoltà siamo obbligati dalla nostra Costituzione non a spingere verso la guerra, bensì verso la sua riduzione, la riduzione del danno continua. Verrò ora a parlare un momento della situazione in Afghanistan. Un paio di giorni dopo l'attentato alle Torri Gemelle, un'Associazione della quale sono una delle portavoce (e che ha un nome più lungo delle sue componenti, essendo una piccola cosa), che si chiama Convenzione permanente di donne contro le guerre, emise un comunicato che naturalmente la stampa trascurò, ma che a noi è molto caro: dicevamo immediatamente che guerra e terrorismo sono crimini contro l'umanità, ambedue; non si elidono, ma si fomentano e pensare di spegnere il terrorismo con la guerra è come pensare di spegnere un incendio con la benzina: una pura follia. Questa motivazione sarei contenta che fosse stata sbagliata, perché a quest'ora ne saremmo usciti, e invece risulta giusta, tanto che anche chi appoggiò con piena coscienza - non ho motivo di dubitarne, fino a prova contraria

che dopo la Seconda guerra mondiale nessun esercito regolare ha mai più vinto una guerra: non gli americani in Corea, non i francesi in Indocina, poi di nuovo gli americani in Vietnam, poi di nuovo i francesi in Algeria, poi i sovietici in Afghanistan, poi persino l'esercito di Israele, così motivato, importante e così sorretto da appoggi internazionali non riesce a venire a capo di un popolo senza terra come i Palestinesi. E anche non mi si dirà che padre e figlio Bush abbiano avuto grandi successi militari, nonostante l'enorme sperpero di mezzi e di vite umane che hanno fatto. C'è qualcosa che non funziona. A me capita di dire (so che non è scientificamente attendibile, ma serve per comunicare) che la guerra è diventata una mastodontica residualità, perché non risolve più i problemi che pone. Può essere ridotta, tenuta sempre sotto controllo e diventare una componente di una scelta politica e diplomatica. Questa è la ragione per la quale è così importante la scelta, la proposta, il tentativo

ma quale scelta non lo è in questo momento? Siamo davanti ad una situazione ancipite, ambigua; siamo davanti a Giano: la pace e la guerra sono lì, davanti al Dio bifronte. E in questo punto qualunque scelta è rischiosa, è rischioso anche scegliere la coazione a ripetere l'aumento della guerra, il suo avanzamento. Questo rischio, però, si sa già che finisce male:

corso, che ci porta, nonostante tutte le nostre piccolezze e piccinerie, un po' al di sopra della situazione così asfissiante in cui spesso viviamo. Diciamo pure che siamo inferiori all'importanza della situazione in cui viviamo: soltanto la prospettiva di una scelta così, se volete, rischiosa, ma volta verso il futuro merita di essere vissuta. Questa è la ragione fondamentale per la quale voteremo «sì»! Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori. Dall'8 marzo, quando il decreto-legge di rifinanziamento delle missioni di pace è stato votato alla Camera, lo scenario internazionale, specie in Afghanistan, è mutato. Non solo, anche in Libano la situazione si è deteriorata. Nel Sud dell'Afghanistan è in corso la cosiddetta campagna di primavera dei talebani, che mirano a riconquistare il potere nel tentativo di distruggere sul nascere la democrazia che si sta cercando di costruire. Una situazione che espone i nostri soldati, come ha sostenuto lo stesso ministro degli esteri D'Alema, a pericoli nuovi e gravi. Le dichiarazioni del Ministro degli esteri di alcuni giorni fa meritavano a nostro avviso una modifica del decreto; visto che questa non c'è stata siamo stati costretti a modificare il voto che avevamo espresso alla Camera. A seguito, inoltre, delle vicende del rapimento del giornalista Mastrogiacomo e delle modalità che hanno portato al suo rilascio si è determinata una crisi nei rapporti con alcuni Paesi alleati nella NATO Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Olanda - che non ha riscontri nel passato. Si è determinato un isolamento dell'Italia anche in Europa, un fatto davvero mai accaduto in termini così pesanti. Una crisi che ha inferto un colpo durissimo alla credibilità e all'affidabilità dell'Italia. Trovo quindi fuori luogo e gratuite talune prese di posizione del presidente del consiglio Prodi e del ministro D'Alema. Il primo prova a fare orecchie da mercante, fa finta che nel frattempo non sia accaduto nulla, e dichiara candidamente di non capire perché si prenda in considerazione la possibilità di non votare il rifinanziamento, visto che il decreto è identico a quello votato alla Camera. Prodi ci ha anche accusato di irresponsabilità; chissà se continua a pensarlo anche dopo le parole chiare dei vertici militari, in particolare del generale Satta, che chiedono un rafforzamento dell'equipaggiamento, nonché un aumento del nostro contingente per far fronte alle mutate condizioni che si sono determinate nei territori afgani sottoposti a controllo italiano. Chi è responsabile allora? Noi che vogliamo mettere i nostro soldati al sicuro e in condizioni di operare al meglio o il Presidente del Consiglio, che per restare incollato alla sedia di Palazzo Chigi volta lo sguardo dall'altra parte, infischiandosi delle loro richieste e pensando piuttosto a soddisfare all'infinito le pressioni della sinistra radicale? Dal canto suo, l'onorevole D'Alema, incapace di un minimo di autocritica - ce lo consenta, onorevole Ministro - ha attaccato dalle colonne di un importante giornale il centrodestra, reo, a suo dire, di voler piegare le scelte di politica internazionale a quelle interne. Onorevole D'Alema, peraltro, lei non si è reso conto di contraddire, in modo palese, le aperture più equilibrate del segretario del suo partito, l'onorevole Fassino, disponibile a rivedere le regole di ingaggio e a dotare i nostri militari di maggiori mezzi per la loro sicurezza. In sintesi, il ministro D'Alema afferma che le regole di ingaggio non si possono cambiare; il segretario del suo partito, onorevole Fassino, siete disponibili a confrontarvi e a cambiare le regole di ingaggio. Respingiamo quindi sia l'atteggiamento evasivo e irresponsabile di Prodi, per il quale nulla è cambiato, sia gli attacchi del ministro D'Alema, al quale ricordiamo che se c'è una coalizione che ha piegato finora le decisioni di politica internazionale agli interessi interni questa è certamente l'Unione, dove è finora prevalso il protagonismo della sinistra radicale. Quella sinistra del presidente onorevole Bertinotti che non ha esitato a parlare di orgoglio nazionale per quanto è stato fatto in occasione della liberazione di Mastrogiacomo e lo ha fatto nel momento di più forte tensione con i maggiori alleati, ossia USA e Gran Bretagna. Noi, diversamente da Bertinotti, non riteniamo che la vicenda della liberazione di Mastrogiacomo, per la quale abbiamo gioito, e in particolare la scarcerazione di cinque o forse più terroristi pericolosissimi, possa essere ascritta nell'ambito dell'orgoglio nazionale, a meno che Bertinotti non pensi, insieme ai suoi compagni, che l'Italia debba iniziare un percorso che porti all'uscita dall'Alleanza Atlantica, che è un vecchio cavallo di battaglia dei comunisti. Una scelta, questa fuori dal tempo e dalle cose. Negli ultimi venti giorni, dunque, abbiamo assistito ad un radicale mutamento della situazione afghana, anche alla luce delle previsioni non rassicuranti sulla campagna di guerriglia scatenata dai talebani, tanto che lei, onorevole Ministro, in più occasioni ha messo in guardia sui pericoli crescenti che i nostri militari corrono quotidianamente. E già indizi concreti si sono avuti con il ferimento di un nostro militare e un agguato ad un nostro mezzo, per fortuna senza gravi conseguenze. Allora bisogna subito sgombrare il campo dalle falsità che a iosa vengono lanciate dalla sinistra contro la nostra posizione critica sulle mancate scelte del Governo. Noi non vogliamo abbandonare i nostri militari, e non lo faremo; vogliamo piuttosto assicurare loro condizioni di maggiore sicurezza, dotandoli di ogni mezzo necessario per resistere agli attentati e agli attacchi che incombono contro di loro. Ma vogliamo anche che i nostri militari, se chiamati a svolgere compiti più impegnativi su richiesta - lo sottolineo, su richiesta - NATO e ONU, siano pronti a farlo. Assumersi un ruolo più oneroso sarebbe un segno di responsabilità corrispondente al peso che un Paese come il nostro deve avere nell'Alleanza atlantica. Ciò non significa che vogliamo fare la guerra ad ogni costo, significa invece che in invece che in un contesto bellico, qual è quello che si vede oggi nel Sud dell'Afghanistan, i nostri militari non possono essere sostenuti da regole che li autorizzino, qualora le circostanze lo richiedessero, ad agire di conseguenza. Ecco perché abbiamo deciso di chiedere modifiche al decreto che voi non avete accettato. Di fronte alla nostra ferma e motivata richiesta di modificare e migliorare il decreto, il Governo e l'Unione hanno risposto con un'irresponsabile chiusura, con la blindatura del provvedimento che si traduce in un «prendere o lasciare», nonostante ci siano i tempi e le condizioni per una terza lettura del decreto alla Camera. Ebbene, signori del Governo, stavolta noi pensiamo che il senso di responsabilità ci debba spingere ancora una volta verso la tutela dei nostri militari. I militari, visti i fatti nuovi di questi ultimi giorni, possono non essere messi nelle condizioni ottimali di intervenire. Ed allora preferiamo astenerci, non possiamo assumerci una responsabilità così grave. Desidero, infine, smentire in Aula un'altra falsità, che il presidente Prodi, e non solo lui, lancia senza provare vergogna: dovesse essere bocciato - sostengono da sinistra - i militari dovrebbero rientrare domani in Italia. È una sciocchezza che fa solo sorridere. Si sappia che questa possibilità non c'è, sia perché i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia

di necessità ed urgenza, un Governo, anche dimissionario, può approvare un altro decreto e le Camere possono approvarlo in tempi rapidissimi. Onorevole ministro D'Alema, fra pochi minuti andremo al voto. Non ci saranno i 158 voti che dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltato. Ci saranno i voti di alcuni senatori a vita, che - ho detto tante volte in quest'Aula - hanno il diritto di votare, ma non hanno vincolo di mandato, vincolo di mandato, e i voti del Gruppo dell'UDC, che mi pare, dalla dichiarazione di voto ascoltata, è un voto dell'emergenza, cioè un voto solo per questo provvedimento. molto probabilmente, onorevole D'Alema, giovedì o venerdì, quando voteremo il decreto sulle liberalizzazioni noi avremo un'altra maggioranza. Questo Governo, Questo Governo, per continuare a governare, un giorno conta i voti degli estremisti di sinistra, come Bulgarelli, Rossi e Turigliatto, e il giorno dopo, sempre per continuare a

visto che ha maggioranze alternative e maggioranze su posizioni politiche estremamente diverse.

Abbiamo chiesto al Presidente di un Governo, per il cui sostegno abbiamo inviato le truppe, di inchinarsi alle esigenze dei talebani

al quale invia i propri militari di abiurare la propria autonomia, la propria autorevolezza, il proprio prestigio scarcerando ben cinque terroristi da esso catturati.

in pochi giorni. Ciò dà il senso del cambiamento del tipo di missione militare che si sta svolgendo in Afghanistan. È cambiato il clima, è cambiato lo scenario politico, mentre il nostro Paese e le nostre truppe sono sempre più isolate, sia a livello politico che territoriale, con mezzi di difesa che le pongono in posizione di subordinazione rispetto ad altri alleati. Abbiamo preso atto in questi giorni di una posizione del nostro Governo che, sulla politica estera, ha accentuato i propri temi su antiatlantismo, su antioccidentalismo, su antiamericanismo sino al punto da ipotizzare che intorno al tavolo della conferenza di pace, della quale si parla, possano sedere addirittura i talebani. Abbiamo assistito dei quali i quali i Presidenti delle più alte cariche istituzionali, del Parlamento in particolar modo, hanno gioito per la diplomazia dei movimenti e non per la diplomazia dei nostri corpi diplomatici o per l'attivismo di quell'apparato dei servizi che, in passato, hanno dato grandi risultati ottenendo la liberazione di nostri ostaggi. Su di essi oggi registriamo, con continuità, il forte,

Siamo dell'idea - ne siamo ancora più convinti dopo la bocciatura del nostro ordine del giorno - che la sicurezza dei nostri militari debba passare per un'assunzione di responsabilità parlamentare, governativa e politica,

siano meglio attrezzati rispetto alle truppe in Afghanistan. In Libano non si spara, in Afghanistan sì. Ci sono gli attentati; è inconcepibile un livello di dotazione di sicurezza inferiore rispetto al Libano. Pertanto, ci siamo attivati. Abbiamo chiesto in quest'Aula una modifica del decreto. Sapevamo che era difficile; l'abbiamo fatto per coerenza politica, ma abbiamo accusato un no da parte del Governo. Abbiamo ricevuto una disponibilità vaga da parte del ministro D'Alema ad accettare l'approvazione di un ordine del giorno che costituisce una dichiarazione di intenti, impegnando il Governo a fare il possibile affinché i nostri militari possano essere salvaguardati e godere una migliore tutela. Ma era soltanto una dichiarazione di intenti, perché quando si è trattato di votare l'ordine del giorno dell'intera opposizione, appoggiato anche dall'alleato UDC, che ha deciso di convergere su questa richiesta, ritenendola

perché se non lo fosse stata avreste potuto votare con noi quella richiesta e quell'ordine del giorno. Invece, vi siete divisi su due temi due temi estremamente delicati che ponevano tematiche attuali e politicamente rilevanti, quali l'esigenza

vi siete divisi su un altro ordine del giorno che postulava l'inammissibilità della conferenza di pace che ammettesse al tavolo i talebani. Anche in quest'occasione

esame che rifinanzia le nostre missioni di pace all'estero. Lo facciamo in piena consapevolezza, sapendo così di manifestare un forte dissenso alla politica estera di questo Governo, che contestiamo e che ci ha portato sempre più a un isolamento internazionale. Lo facciamo anche per dare un segnale al Paese e al Governo: faccia in modo, assumendosene la piena responsabilità, di tutelare bene e meglio i nostri militari che abbiamo mandato consapevolmente lì a rischiare la vita.

le vicende di questi giorni e le discussioni che le hanno accompagnate hanno rafforzato in noi la convinzione di votare a favore del provvedimento di rifinanziamento delle 22 missioni internazionali che impegnano in 18 Paesi più di 8.000 militari italiani, oltre ad alcuni civili; tutti impegnati in delicati teatri di crisi dove, con le loro capacità professionali, con il loro spirito d'umanità, con un'attenzione unica alle popolazioni civili, stanno mettendo al servizio della pace quelle virtù riconosciute e apprezzate da tutti. Noi non ci stancheremo mai di ringraziarli per quello che stanno facendo. Ci fanno sentire orgogliosi di essere italiani. E non si possono dimenticare in questa circostanza anche quanti hanno perso la vita. Noi abbiamo già potuto misurare quanto sia pericoloso operare in quelle zone, da ultimo, nelle terribili ore del sequestro di Mastrogiacomo. Siamo contenti di aver salvato la sua vita, tanto quanto siamo addolorati per la morte atroce del suo autista; così come stiamo seguendo con ansia gli sviluppi della vicenda che riguarda il suo interprete e il dirigente dell'ospedale di Emergency. Sono stati giorni e situazioni molto difficili per tutti. Qui vogliamo confermare al Governo tutto il nostro apprezzamento per come è stata gestita la vicenda. Credetemi, cari colleghi, consideriamo del tutto privi di fondamento quei rilievi critici postumi che abbiamo ascoltato, chiaramente strumentali e finalizzati - come è stato anche ammesso nei vostri interventi - soltanto a sostenere la decisione di cambiare il voto in quest'Aula. Fornire ai nostri militari il sostegno necessario per portare avanti quei difficili compiti noi lo riteniamo un dovere, prima ancora che un atto di responsabilità. Tutti, le forze politiche di maggioranza e di opposizione, siamo chiamati ad una prova di coerenza. Sono missioni che in questo Parlamento, caro collega Schifani, abbiamo già discusso e approvato a larghissima maggioranza, indipendentemente dal colore dei Governi che in questi anni si sono succeduti. C'è davvero qualcosa di paradossale nel vostro comportamento, in chi ha predicato la necessità della lotta al terrorismo al fianco degli alleati e che oggi sembra considerare quella necessità una variabile dipendente, rispetto ad esigenze di politica interna, subordinando il voto sulle nostre missioni a valutazioni di tattiche parlamentari, Gruppi Ulivo e RC-SE).* È incomprensibile, è inaccettabile. Nei giorni scorsi qualcuno ha anche provato a spiegarci che in questi mesi il comportamento del Governo ha fatto perdere credibilità all'Italia. A parte il fatto che noi non crediamo che si possa considerare perdita di credibilità la determinazione con cui si difendono le prerogative di un Paese, per esempio di fronte ad improvvide ingerenze di alcuni ambasciatori, non si perda credibilità se si pretende dai Paesi alleati, e nella fattispecie dagli alleati Stati Uniti, una cooperazione giudiziaria perché si faccia piena luce sulla morte di un nostro eroe, servitore dello Stato, come Nicola Calipari. Un Governo responsabile sa tenere fede alle alleanze internazionali, sa rispettare gli impegni, senza mai rinunciare a difendere l'orgoglio e la dignità nazionali. Questa nostra condotta, secondo me, ha aumentato la credibilità dell'Italia e lo dimostra l'attenzione e il rispetto con i quali ci hanno risposto anche in queste ore dal Dipartimento di Stato. Semmai un colpo mortale alla nostra credibilità verrebbe dalla mancata conversione di questo decreto. E la maggioranza di quest'Aula, il voto dei senatori della maggioranza e di quelli del Gruppo UDC, consentiranno di tenere ancora alta la credibilità internazionale dell'Italia. Una credibilità indispensabile per consentire il buon esito delle missioni in cui siamo impegnati, a partire da quella in Libano, che ha segnato una svolta nella vicenda internazionale, laddove sono tornate protagoniste le Nazioni Unite, di cui sembrava non vi fosse più bisogno. Noi possiamo sentirci tutti - dico tutti - orgogliosi di aver consentito all'Italia di svolgere un ruolo cruciale nel favorire l'invio e, ora, nel guidare una forza multinazionale con europei, turchi, indonesiani, soldati del Qatar, insieme cristiani e musulmani, che lì hanno fermato una guerra e ora presidiano la pace, con lo stesso spirito con il quale siamo presenti nei Balcani, nel Darfur o in Afghanistan. Certo, quest'ultima missione richiama più di ogni altra l'attenzione per i rischi che oggi si paventano, per la dimensione della nostra presenza militare, ma anche perché quello è uno snodo nevralgico dal punto di vista geopolitico, collocazione: un crocevia tra le vecchie e le nuove potenze del mondo globale. Da sempre l'Afghanistan è una delle porte tra Oriente ed Occidente, che riflette la complessità del nascente multipolarismo. Non è un caso che, fin dai tempi del «grande gioco» ottocentesco, chiunque si sia cimentato con quella situazione, senza tenere conto di quanto complesso fosse quello scenario, ha avuto vita difficile e ha registrato amare sconfitte. Deriva anche da questa esperienza storica, oltre che dalla presa d'atto di una situazione che rischia di degenerare, la consapevolezza che non basta la presenza militare, che occorre l'iniziativa politica. Oggi la presenza militare della NATO, sotto il mandato delle Nazioni Unite, resta a nostro avviso indispensabile e in questo quadro va confermata la nostra missione. Siamo confortati, caro Ministro, dalle rassicurazioni, che anche qui ci sono state fornite, circa la piena disponibilità a valutare positivamente tutte le esigenze, informando il Parlamento, per garantire la protezione dei nostri militari e il pieno espletamento della missione. Ma non basta. La presenza militare non basta. Di qui nasce la nostra richiesta di una conferenza internazionale di pace. di pace. Non è un contentino a nessuno ed è impressionante la superficialità che traspare da questa argomentazione. Io consiglierei di leggere la proposta di conferenza internazionale presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazione Unite. Si potrà constatare che è una proposta seria, non molto diversa da quella del tavolo regionale che si è finalmente aperto sull'Iraq, e che deve vedere protagonisti, con il Governo afghano, i Paesi confinanti, a iniziare dal Pakistan, oltre ad Iran, Cina, Russia, India e quei Paesi e quelle organizzazioni che sono impegnate nell'area. una proposta impegnativa sulla quale occorrerà ancora lavorare, ma che fa registrare già i primi apprezzamenti. in tanto possiamo sostenere questa iniziativa in quanto sappiamo assumerci le nostre responsabilità. Quando si è all'opposizione, contro la guerra si fanno i cortei; quando si è al Governo, contro la guerra bisogna agire concretamente. Noi lo stiamo facendo. Noi lo stiamo facendo. È triste constatare come un passaggio così importante della vita del Paese sia vissuto da alcune forze parlamentari con assoluto tatticismo; una logica che mortifica il principio di responsabilità, ma, soprattutto, sancisce il rifiuto della nozione di interesse nazionale, che è l'unico superiore interesse nel nome del quale noi voteremo a favore di questo provvedimento. Lo dobbiamo ai nostri militari, lo dobbiamo all'Italia.

il nostro Paese avrebbe bisogno di una politica estera lineare, credibile e condivisa; una politica che vada oltre le logiche rigide degli schieramenti e le asfittiche congiunture parlamentari e realizzi i concreti interessi della nostra comunità; una politica che deve possedere un respiro strategico, che abbia l'ambizione di superare la stagione di un Governo e addirittura le cadenze delle legislature per offrirsi quale interlocutore affidabile alla comunità internazionale. Una politica estera che abbia come baricentro il Mediterraneo, in cui dispiegare il ruolo plausibile di potenza regionale impegnata, in un quadro multilaterale, nella stabilizzazione dell'area attraverso la lotta al terrorismo; che operi per disinnescare i conflitti regionali attuali e potenziali attraverso una seria politica di cooperazione allo sviluppo che può rappresentare anche una grande opportunità economica per aree importanti del nostro Paese proiettate in questo contesto geografico e culturale. Per questo occorrerebbe una classe dirigente consapevole delle proprie responsabilità, che voglia sfuggire alle tentazioni del tatticismo e della strumentalità per individuare le opportune convergenze attorno al nucleo inscindibile dell'interesse nazionale. invece, partecipando a questo dibattito preceduto da un'attesa spasmodica, abbiamo assistito al solito sterile canovaccio: da una parte, un Governo avvinghiato alla sua fragile maggioranza e costretto da questa a ribadire posizioni minime, rigide ed asfittiche che hanno solo l'obiettivo di garantirne l'esistenza in vita, qualunque essa sia; dall'altra, un'opposizione per certi versi schizofrenica che, trascinata dal sogno della spallata ad ogni costo, sbanda troppo spesso contraddicendo sé stessa, i suoi princìpi ispiratori e perfino il voto espresso positivamente sul medesimo provvedimento pochi giorni fa nell'altro ramo del Parlamento. conferma così nella pubblica opinione, sempre di più, lo sconcerto e la profonda sfiducia nella capacità di questo sistema politico di saper assicurare il benessere delle comunità al di là degli interessi particolari degli schieramenti cui si appartiene. Il Movimento per l'Autonomia, nella sua autonomia, non rintracciando in alcuna delle posizioni espresse la completa realizzazione degli interessi della nostra comunità nazionale, dichiara la propria insoddisfazione per questo contesto politico che produce tali esiti e rende esplicito il proprio dissenso e la propria distanza da questo sterile rituale abbandonando l'Aula e non partecipando alla votazione.